Presidente, la giornata di ieri si è conclusa con l'auspicio, da parte delle opposizioni, di poter avere un momento di riflessione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi perché ci auguriamo di non dover vivere un'altra giornata come quella. Nell'economia dei lavori - lo dico al presidente Malan, al presidente Romeo e al presidente Gasparri

Invece, siccome si è applicata la regola del canguro, mettendo in votazione in alcuni casi una parte

più di un terzo degli emendamenti previsti non ci sono più. È evidente che, siccome abbiamo tutto l'impianto della proposta di riforma che noi avversiamo e contestiamo, ma che dobbiamo affrontare pezzo per pezzo in quest'Aula, signora Presidente, penso che sia necessaria e urgente la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché riteniamo che non si possa proseguire nei nostri lavori così come abbiamo fatto ieri, semplicemente perché rischiamo di ritrovarci di nuovo nella condizione di uno scontro, prima di metodo e poi verbale, e vorremmo evitarlo. Ovviamente, se ci dovessero essere forzature,

Malan, ma solo una valutazione del quadro generale. Stiamo chiedendo regole trasparenti e penso che siano dovute. Non è in discussione l'utilizzo del canguro, perché ieri mi sono sentito rispondere dal presidente La Russa che si faceva anche prima. Qui il tema non è l'utilizzo di tale strumento, ma quando si utilizza e per cosa. Tutto questo va definito prima

già ribadito ieri alla fine della seduta, aggiungo un elemento. Vi sono state delle legittime scelte della Presidenza rispetto ad emendamenti verso i quali è sospeso il giudizio di proponibilità del testo, e in più è stata accantonata una parte di un emendamento che riprende, anche se in maniera meno ampia, un emendamento ancora da discutere per una decisione politica, per un approfondimento di merito su quel testo. Stiamo parlando di una riforma importante, verso la quale sono chiare le posizioni politiche, ma di certo maggioranza e opposizione condividono che sia una riforma che incide profondamente sulla Costituzione, secondo noi in modo negativo, secondo maggioranza e Governo in modo positivo. Sicuramente è una riforma molto incisiva della nostra Costituzione.

Ritengo che una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi debba essere fatta prima di ricominciare a votare, altrimenti potremmo incorrere nella condizione di perdere per strada dei pezzi che magari hanno rilevanza, o per le opposizioni, o anche per ragionamenti della maggioranza. assieme al presidente Boccia, ma penso anche assieme agli altri Presidenti dei Gruppi di opposizione, che non si ricominci fino a quando non venga fatta chiarezza in sede di Conferenza dei Capigruppo, che credo possa agevolare il lavoro e non certamente con spirito, in questo caso, ostruzionistico. io parlo a nome di un Gruppo che ha presentato soltanto 14 emendamenti, come abbiamo già avuto occasione di dire, non un Gruppo votato a un ostruzionismo estremo. Come la ministra Alberti Casellati sa bene, noi siamo aperti all'idea di una riforma, anzi pensiamo che una riforma sia indispensabile; l'importante naturalmente è scriverla bene. proprio per esperienza personale, avendo io frequentato queste Aule da Sottosegretario alle riforme costituzionali negli anni 2014-2016, penso che sia interesse di tutti che questo percorso di riforma costituzionale vada avanti con un'Assemblea gestita nel modo più pacato possibile, seppur ovviamente con il calore degli argomenti e con la passione politica che risvegliano riforme così importanti. Penso che sia nell'interesse anche del Governo, della ministra Alberti Casellati, del relatore Balboni e del presidente Malan non esacerbare gli animi. Sia Sia nelle repliche del relatore e della Ministra che negli interventi della Presidenza di ieri, io francamente, lo dico da ex Sottosegretario alle riforme, avrei provato a tenere un ambiente un po' più tranquillo. Penso che l'onere della della gestione dell'Aula e della gestione di un processo più collaborativo stia sulle spalle di chi ha interesse a portare avanti questa riforma. In questo quadro, il mio e il nostro incoraggiamento alla maggioranza e al Governo è, tra le altre cose, quello di chiarire il quadro delle regole e il campo di gioco che ci stiamo dando per questa riforma, con trasparenza e soprattutto in anticipo. Anch'io ho trovato poco avveduta la mossa del presidente La Russa di prendere una decisione senza socializzarla con i Capigruppo, perché è chiaro che poi questo solleva una reazione comprensibile. Se si riuscisse a convocare una Conferenza dei Capigruppo regolamentare, in un certo senso, rispetto a questo particolare disegno di legge, io credo che ciò contribuirebbe moltissimo a una gestione dell'Aula e del processo di riforma più tranquilla e più collaborativa, che - ripeto - secondo me è un onere e un interesse soprattutto dei proponenti di questa riforma. A me pare che una Conferenza dei Capigruppo, da convocare il più presto possibile, sia un'idea eccellente, proprio per una questione di chiarezza e di trasparenza, ferme restando la chiarezza e la trasparenza delle posizioni che in quest'Aula sono state rappresentate in modo molto evidente (è chiaro che ci sono delle differenze di opinione). Penso che questo passaggio sarebbe molto utile, molto costruttivo e molto proficuo. Quindi, pur rappresentando un Gruppo che di questi 3.000 emendamenti ne ha presentati soltanto 14 e che non è pregiudizialmente contrario all'idea che le riforme costituzionali in questo Paese si facciano, perché secondo noi sono indispensabili, credo anche che un ordinato processo legislativo sia importante. Mi permetto di dire, sempre sulla base dell'esperienza precedente, che ieri siamo partiti nel peggiore dei modi. Quindi, se riusciamo in corsa a rimettere l'automobile in carreggiata, credo che sarà meglio per tutti.

Noi ovviamente abbiamo rivendicato e rivendichiamo il fatto di aver presentato emendamenti anche ostruzionistici, però chiederei che, prima di continuare questa discussione, sia chiaro

le procedure; se sono chiare le procedure, ognuno ovviamente si comporta di conseguenza, anche perché - lo dico per me non diamo un bello spettacolo se c'è confusione e se la discussione in Parlamento si trasforma più o meno in una rissa, come ieri in qualche occasione è accaduto. Sottolineo quindi la richiesta di avere chiaro come si procede. Per questa ragione,

Presidente, ritengo assolutamente comprensibile la richiesta di una Conferenza dei Capigruppo, che immagino poi la Presidenza convocherà quando lo riterrà (sicuramente in giornata); dopodiché, rispetto ad alcune considerazioni fatte e anche di fronte a una serie di interventi reiterati, ieri non ho fatto alcuna osservazione, però colgo l'occasione per fare un ragionamento sulle regole, che alcuni richiamano ai fini delle votazioni degli emendamenti. Arriviamo a votare in Aula questo provvedimento al ventesimo mese della legislatura. È un provvedimento che riguarda l'elezione diretta del *Premier*, che noi avremmo voluto declinare anche in forme diverse, come il presidenzialismo, già questo disegno di legge rappresenta una forma di apertura a tesi diverse. Nel corso del dibattito, dovendo fare molti interventi ostruzionistici, si rischia di ripetere anche cose non vere:

questo tema fa parte delle priorità programmatiche della coalizione di centrodestra, che ha vinto le elezioni e ha la maggioranza in Parlamento, quindi non deve fare alcuna vessazione, ma non può nemmeno essere paralizzata. L'opposizione infatti si deve opporre, ma non paralizzare i lavori o trasformarsi in maggioranza. Lo abbiamo imparato tutti, perché a rotazione i ruoli cambiano secondo gli esiti elettorali, quindi non è che a noi non sia capitato di vederci cangurati, contingentati o bloccati da fiducie. Insomma, lo sappiamo tutti, altrimenti poi si racconta

di darci da fare, mentre non trovo nessuno che mi dica che stiamo correndo troppo. Non so se a lei qualcuno contesti la fretta al ventesimo mese di legislatura: a me contestano il contrario. Ieri abbiamo discusso a lungo anche dei senatori a vita: non è questa l'occasione per entrare nel merito, ma mi avrebbe fatto piacere confrontarmi col senatore Piano, che ho visto un paio di volte in quest'Aula, anche in occasioni molto politiche (venne a votare la decadenza di Berlusconi; è venuto un'altra volta a farci una lezione sul rammendo dell'Italia;

ne ho conosciuti meno del presidente La Russa, che è più grande di me e ha detto di averne conosciuti molti, però in quest'Aula ho incrociato Cossiga e Andreotti, abbiamo fatto anche interventi celebrativi, quando questi Padri della Patria; ricordo il novantesimo compleanno di Andreotti, che sentiva i nostri interventi infastidito, perché si rendeva conto che il tempo scorreva. Ho fatto una riflessione e lo dico al senatore Franceschini, che vedo qui: in quell'elenco importantissimo, l'area politico-culturale che ha governato questo Paese per una decina d'anni non trova nessuna personalità che sia stata nominata

Conferenza dei Capigruppo e dico che il Regolamento è ampio e consente molto: non è che mi meravigli dell'ostruzionismo, perché tale è e fa parte della logica della democrazia e della dialettica; meno male che siamo un Paese libero, in cui si può fare ostruzionismo, ma tale è.

la Presidenza seguirà le regole. Il Presidente e i Vice Presidenti sanno bene cosa si deve fare. Dopodiché, ci sono tante altre previsioni nei regolamenti: c'è il contingentamento dei tempi, c'è la possibilità di prendere una decisione. Lo dico al presidente Boccia, che ogni tanto chiede cosa ne penso. Noi abbiamo il diritto di decidere. L'opposizione si può opporre, ma non può impedire alla maggioranza di esercitare il mandato democratico che ci hanno affidato gli elettori. E noi intendiamo esercitare il mandato democratico che ci hanno affidato affidato gli elettori. Quindi, non ci possono essere imposizioni da parte nostra e non ci possono essere impedimenti a legiferare da parte vostra. La Conferenza dei Capigruppo ci darà le linee direttive. Stiamo, giustamente, assistendo a questi interventi che, lo ripeto, sono legittimi. Non crediate, però, che si impedisca di attuare un programma elettorale di democrazia diretta. C'è chi vuole che i capi del Governo li scelga il palazzo; il centrodestra e, quindi anche Forza Italia, vuole che i capi del Governo li scelga il popolo. E noi vinceremo questa grande battaglia di democrazia e di partecipazione.

Parlando della richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, ricordo che abbiamo tutti concordato che si sarebbe lavorato dalle ore 9 anziché dall'ora consueta per poter andare avanti con i lavori, dando spazio ai numerosi interventi, in grande maggioranza dell'opposizione, come è anche normale in una situazione di questo genere. Duecento più cinque senatori sono stati convocati stamattina alle 9, non per aspettare, durante la sospensione, dovuta alla Conferenza dei Capigruppo, ma per andare avanti nei lavori. Questo era quanto era stato concordato.

in assoluta aderenza alla realtà. Sono trent'anni che si usa questo metodo. In particolare, ricordo, da qualcosa più degli ultimi vent'anni e mai è stata fatta questa richiesta, anche perché è sotto gli occhi di tutti e si sa benissimo come funziona quando ci sono degli emendamenti che iniziano allo stesso modo e questa prima parte è tale da avere una qualche forma di senso compiuto, la si vota; se respinta, la seconda parte decade. Per cui, se si vuole votare la seconda parte, si vota a favore È stato sempre fatto così. Mi permetto di ricordare quanto ho già detto ieri. Due legislature fa, quando erano presenti ventisette senatori dell'attuale opposizione consenzienti con quel metodo, vi furono numerose richieste di voto segreto, perché congrue rispetto al Regolamento. Esse furono molto limitatamente accolte dalla Presidenza. Poi, però, col metodo del canguro anche quei pochissimi emendamenti su cui era stata accettata la richiesta di votazione a scrutinio segreto

Detto questo, i meccanismi sono ben noti. Per convocare una Conferenza dei Capigruppo, credo che ci sia ampiamente spazio per farlo più tardi, e penso che dovremmo andare avanti con i nostri lavori.

numerosi interventi, più che legittimi nel loro numero e anche nel loro contenuto, in molti dei quali sono arrivati epiteti anche pesanti, per non dire insulti, è anche normale che, nel

della Conferenza dei Capigruppo è una questione già emersa nel corso della seduta di ieri, pertanto la Presidenza ha già fatto pervenire la sua posizione, che riassumerei

siamo sempre sull'articolo 1 e siamo sempre qui a fare dei tentativi di rimediare a una riforma che si sta presentando sempre più disastrosa, con conseguenze nefaste per il Paese. Vorrei però fare con voi una riflessione. È una riforma che teoricamente riguarda l'elezione diretta del *Premier*, così viene presentata, e il primo articolo non parla dell'elezione diretta del *Premier*.

da ciò che c'è scritto realmente. Questi *slogan* e queste modalità di presentare la riforma stanno nascondendo la verità; stanno dando l'illusione che si tratti solo di scegliere quella figura istituzionale che già conosciamo, mentre sapete benissimo che non è così. Sapete benissimo che state cambiando e rafforzando quei poteri.

Pensate ad esempio alle opere di Freud sulla psicologia delle masse; pensate a Le Bon sulla psicologia delle folle o a Elias Canetti. folle o a Elias Canetti. Non so se lo si sta facendo apposta oppure no, però fateci caso, gli elementi sono sempre gli stessi. Si parte intanto dalla paura; finta o vera che sia, si crea la paura. Abbiamo sentito Giorgia Meloni e il ministro Alberti Casellati: questa instabilità del Governo ci impoverisce, è il problema economico del Paese. Questa è la paura. Non si dice però che in realtà i problemi sono altri; sappiamo che abbiamo un problema democratico, che non è quello di rafforzare l'Esecutivo, ma semmai il Parlamento. Non tenete conto che il problema più grande per esempio è la corruzione, contro la quale non mi sembra che voi stiate facendo granché. Il MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura ha fatto un provvedimento per contrastarla e l'Europa ci ha riconosciuto un grande passo in avanti nella lotta contro la corruzione. Voi invece spuntate le armi alle procure, cercando di indebolirle, per per assecondare un capriccio di una parte politica. Quindi state creando un problema maggiore di quello che volete risolvere dal punto di vista economico.

riforme, ma i problemi dell'Italia sono altri, non so se ve ne siete accorti: i prezzi al consumo stanno aumentando, i costi degli affitti soltanto qui a Roma stanno raddoppiando, gli stipendi hanno soltanto un valore nominale, non hanno un valore reale: sono una valuta, non un valore; abbiamo bisogno di fare una riforma del lavoro; del lavoro; rifiutandovi di inserire un salario minimo, state legittimando lo sfruttamento dei lavoratori; ci sono aree di crisi industriale complessa che aspettano le vostre risposte; ci sono carenze infrastrutturali. State dicendo che questa è la madre di tutte le riforme, ma tutti i problemi del Paese li conoscete o ve ne siete dimenticati? inoltre, il fatto che poi questa riforma che sta centralizzando il potere sta dimenticando anche l'ascolto dei territori. Su questo tornerò più avanti, perché non credo di avere tempo, però vi faccio notare che abbiamo, ad esempio, le aree sismiche. Questo Governo non si è accorto che ha un suo commissario al sisma che conosce il territorio, eppure voi varate un provvedimento che attua un blocco perché non sono stati adeguati i costi parametrici e un altro provvedimento che poi avete dovuto modificare, perché in esso si eliminava il superbonus che, insieme ai costi parametrici attuali, consentiva la ricostruzione. Avete fatto un provvedimento senza neppure ascoltare un vostro parlamentare che voi avete nominato come commissario.

Signora Presidente, noi abbiamo tante volte chiesto nel corso di questo confronto di capire le ragioni della soppressione della prerogativa, che oggi la Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica, di nominare fino a cinque senatori a vita. Ieri, dopo nostre ripetute sollecitazioni,

siccome il Senato è una assemblea elettiva, allora i senatori nominati dal Presidente della Repubblica - una componente eccentrica, un'anomalia, sono qualcosa che non ha ragione d'essere. Devo dire la verità, con tutto lo sforzo di comprensione possibile, faccio fatica a capire perché si debba far venire meno questa prerogativa del Presidente della Repubblica e questa natura plurale dell'Assemblea del Senato.

di pluralismo politico e sociale. I nostri Costituenti argomentarono, cioè, con una certa solidità la compatibilità tra un'Assemblea espressione del pluralismo politico e sociale e la presenza di figure espressione delle eccellenze e di una di una sensibilità ulteriore e anche con la necessità di avere comunque una presenza che potesse mitigare eventuali conflitti politici che, all'interno delle Assemblee, è per certi aspetti fisiologico che si determinino. Ho quindi cercato di capire quale fosse il vero senso della risposta e devo dire che, a pensarci con più attenzione, forse la risposta è incomprensibile solo perché parziale, solo perché è una risposta che omette quella che in realtà è la vera ragione della scelta della maggioranza. La vera ragione sta in questo: la riforma

direttamente eletta dai cittadini, non più un'Assemblea elettiva espressione del pluralismo politico e sociale, ma espressione dell'elezione del Presidente del Consiglio; cioè una Assemblea, sì, elettiva, ma in conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. Infatti nella riforma si prevede che il Parlamento non sia più composto da deputati e senatori direttamente eletti dai cittadini, come prescrivono gli articoli della Costituzione, ma eletti in conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. Allora, effettivamente, avere una presenza di senatori che non sono eletti in conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio è un'anomalia, un'incoerenza. Se tutti i senatori devono essere espressione

A questo punto mi è più chiara la ragion d'essere di tanta ostilità nei confronti dei senatori a vita e di tanta reticenza nello spiegare il perché si dovrebbe abrogare radicalmente questa presenza anziché, come pure è stato proposto in diversi emendamenti, ragionare su una rimodulazione e su una ridefinizione delle loro prerogative,

tutto il potere in una sola figura e di ridurre l'intera democrazia rappresentativa alla sola scelta del capo, senza più neanche prevedere che le Assemblee esprimano una composizione che non sia appunto diretta conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. Grazie Presidente, lo dico in maniera meno sottile di come ha fatto adesso, secondo me davvero con grande capacità, il senatore Giorgis, con il quale peraltro ci siamo confrontati tante volte in questi mesi in Commissione affari costituzionali come sempre, non foss'altro per il fatto che conosce con particolare dovizia il diritto costituzionale, ci ha spiegato alcuni aspetti che che probabilmente sfuggono a un primo sguardo e che poi invece si rivelano particolarmente corretti e giusti. Quindi lo dico in maniera più rozza di come ha fatto lui ora, cercando però anch'io di focalizzare l'attenzione su questo punto. Se capisco bene, il tema è che noi non possiamo avere, come ci ha spiegato ieri il presidente Balboni quando - bontà sua, e di questo naturalmente lo ringrazio -

Si potrebbe molto discutere su questo, sulla natura elettiva e anche sulla storia del Senato: non tutti sanno che, quando il Senato nacque, un numero abbastanza significativo dei senatori all'epoca non era di natura elettiva, perché subito dopo la fine della dittatura e del fascismo si scelse di nominare una serie di figure che erano state particolari espressioni dell'antifascismo. È un'altra storia, sono altre vicende, che però pure dovrebbero essere approfondite, perché fanno parte della storia di questo Paese.

che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Ieri è stato fatto l'elenco di queste 38 figure, che penso tutti, in maniera unanime,

che sfuggono in maniera sostanziale al principio dell'elettività che viene raccontato, perché sono eletti per trascinamento,

sappiamo bene che quelli che tra di noi sono stati eletti nei collegi uninominali in realtà sono già stati eletti per trascinamento; infatti, per come è fatto l'attuale sistema elettorale, è largamente preponderante il voto alla lista bloccata piuttosto che il voto al collegio. Io sono assolutamente convinto che una larga parte degli elettori che hanno votato alle scorse elezioni politiche nemmeno sapeva dell'esistenza di una contesa nel singolo collegio tra un candidato del centrodestra, uno del centrosinistra, uno del MoVimento 5 Stelle e uno del terzo polo.

e che comporterà, come stiamo cercando di dire da molti mesi a questa parte, in Commissione prima e adesso in Aula, questa cosiddetta elezione a strascico o elezione per trascinamento.

che cinque senatori a vita sfuggono al principio dell'elettività e allora non vanno bene, mentre 110 senatori, che sfuggono clamorosamente al principio dell'elettività, perché sono eletti per trascinamento, rispondono alla volontà del popolo sovrano? A me pare davvero una gigantesca ipocrisia. penso che il punto sollevato dal collega Giorgis sia corretto e vorrei affrontarlo anche da un altro punto di vista. Avendo scelto, con l'impostazione di questa riforma, di eleggere contemporaneamente e in modo consequenziale il Parlamento e il Presidente del Consiglio,

super coerente, forzosamente molto coerente, credo che avere cinque voci completamente fuori dal coro, cinque voci che esprimono un'altra logica, arricchisca in modo essenziale la diversità

per esempio, con alcuni memorabili - storici, mi permetto di dire - interventi della senatrice Segre, come quello che ha dato inizio a questa legislatura) sia importante. Penso che, in particolar modo in quel tipo di Senato

A me sarebbe molto piaciuto utilizzare questa occasione per provare a toccare alcuni aspetti rimasti pendenti dopo la sciagurata riduzione del numero dei parlamentari. avuto occasione di ricordare che, con la riduzione di questo numero, il ruolo dei delegati regionali nell'elezione del Presidente della Repubblica non è più proporzionato.

non mi stupisco perché questo passaggio sulla struttura del Parlamento dentro questa riforma costituzionale era - sì - un'occasione ancora più grande. Desidero

accettabile se fosse stata conseguenza di una revisione organizzativa complessiva del nostro sistema parlamentare. Se una sola Camera desse la fiducia (e io la riporterei addirittura a 630 deputati) potremmo

vita. Credo che, finché siamo in tempo e soprattutto in vista dell'approvazione della legge sull'autonomia differenziata (vedo presente il ministro Calderoli), l'idea di ritornare a pensare a un Senato delle Regioni Regioni vada colta. È questo il momento, perché se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più, nel senso che dovremo aspettare chissà quanti anni. Quindi, visto che siamo in prima lettura e possiamo agire, invito davvero il Governo a riguardare l'emendamento e, se possibile, a esprimere parere favorevole per andare in quella direzione.

senatore Balboni, ha dato anche un'altra spiegazione, dicendo che siamo l'unico Paese in tutto il mondo ad avere i senatori a vita.

esaurienti e penso anch'io che sia una mossa populista. Se dovete affrontare un *referendum*, potete dire che avete

di quelli che hanno studiato, hanno fatto ricerche, magari hanno addirittura vinto un premio Nobel:

C'è anche un altro aspetto per me molto importante. Pensate al ruolo della senatrice Segre, al suo ruolo in questo momento storico in cui l'antisemitismo si

siccome continuo a essere chiamato in causa, vorrei dare alcune risposte ai colleghi. La prima risposta, attraverso lei, Presidente, vorrei darla al senatore De Cristofaro.

sia io che il ministro Alberti Casellati su questo tema siamo intervenuti a più riprese. E ricordo benissimo di avere fornito le stesse spiegazioni che ho dato qui in Aula e anche in Commissione, in occasione, ad esempio, della replica dopo la discussione generale. Mi dispiace che altri colleghi non abbiano abbiano ascoltato nemmeno quello che ho detto in replica qui in Aula l'altro giorno e le spiegazioni che ho dato ieri, o, peggio ancora, le abbiano ascoltate e travisate. punto primo. Non è vero - e l'ho detto anche ieri - che la riforma che vogliamo introdurre col premio di maggioranza alla coalizione che esprimerà il *Premier* eletto provocherà l'elezione di ben 110 senatori per trascinamento. Non è assolutamente così e questo ce lo dice l'aritmetica, ce lo dice la matematica. Se il premio di maggioranza sarà al massimo del 15 ne consegue che il rimanente 85 per cento sarà espressione proporzionale dei voti ricevuti dalle singole forze politiche, o dalle singole coalizioni. Quindi, al massimo il premio sarà del 15 Ma attenzione: al massimo, perché - come ho cercato di spiegare, ma forse il limite è mio - questa riforma avrà inevitabilmente un effetto bipolarizzante, chiaramente le coalizioni saranno costrette a presentarsi nel modo più competitivo possibile. Questa riforma avrà anche un effetto importante per le opposizioni, che non avranno più una ragione, se non esponendosi al pubblico ludibrio, di presentarsi divise in quattro di utilizzare come argomento principale della propria campagna elettorale quello non di proporre un programma alternativo al centrodestra, ma di far vincere il meno possibile l'avversario. Se questo vi sembra un sistema politico al quale aspirare, sinceramente noi la pensiamo diversamente, non nell'interesse di questo o di quello schieramento, bensì nell'interesse della democrazia italiana. Secondo noi, l'unica vera forma di democrazia compiuta - non mi stancherò mai di dirlo - è la democrazia dell'alternanza, la democrazia che si basa su due schieramenti altrettanto competitivi, che offrano un programma di Governo per il Paese e per il futuro. Questa riforma non è fatta per l'oggi. Ce ne siamo accorti anche noi che abbiamo una maggioranza ampia in questo Parlamento e vi ringraziamo di ricordarcelo in continuazione. Ma il problema non è oggi: il problema è domani. Noi vogliamo una democrazia compiuta per questo Paese. È questa la ragione che ispira la nostra riforma. Seconda questione: ci sono altre assemblee elettive nelle quali esistono figure come i senatori a vita? No, cari colleghi. Mi dispiace, senatrice Unterberger. Mi dispiace, senatore Mi dispiace, senatore Scalfarotto. La Camera alta del Regno Unito non è un'assemblea elettiva: è nominata. Quindi è ovvio che, in un'assemblea di nominati, ci siano dei nominati. Non capisco qual è il vostro ragionamento: la Camera dei Lord è un'assemblea di nominati. Mi sono permesso di fare un altro ragionamento, relativo alle assemblee elettive. E allora c'è un'unica assemblea elettiva,

te, lo dico a te, perché l'unico caso al mondo - in cui c'è un'assemblea elettiva che comprende dei senatori a vita - è in Russia, con una riforma voluta da Putin nel 2020. E allora, cari colleghi, io non uso questo come argomento. Io vi dimostro che il vostro argomento è sbagliato, perché in questo caso non vi interessa ci sia l'unico caso al mondo di senatori a vita. Questo non vi interessa. Ma, quando parliamo del *Premier* eletto, improvvisamente vi interessa il confronto. O il confronto con gli altri Parlamenti vale sempre, o il confronto con gli altri Parlamenti non vale mai. Io sono per la seconda: non vale mai. Infatti cosa ho detto? Siccome questa è un'Assemblea elettiva, mi sembra ragionevole che ci si debba entrare con il consenso degli elettori. Mi sembra ragionevole. Ho anche sottolineato che condivido quello che diceva il Partito Comunista Italiano all'Assemblea costituente. Lo so che vi dà fastidio che lo ricordi, ma è così. All'Assemblea costituente il Partito Comunista Italiano sosteneva esattamente questa posizione, e cioè che in un'Assemblea elettiva ci si entri con i voti. Scusate, ma mi sembra democratico. La presenza dei senatori a vita distorce la rappresentanza parlamentare e oggi non trova più alcun motivo di esistere. Lo ha detto il pericoloso sovranista senatore Alberto Balboni? No, lo ha detto e lo ha scritto, in un disegno di legge costituzionale, il senatore Vito Crimi, MoVimento 5 Stelle, attuale consulente del Gruppo, dopo essere stato Capogruppo. Andate a leggere. *(Applausi)*. Ma c'è un ultimo argomento, che è il più importante. Voi state strumentalizzando, cari colleghi, in un modo che non voglio definire, perché lo lascio definire voi, una figura straordinaria come la senatrice Segre, che ha il rispetto e l'ammirazione di tutta quest'Assemblea, dall'estrema sinistra all'estrema destra (estrema certamente alla mia). La state strumentalizzando e non vi rendete conto che state proponendo di trasformarla in una senatrice di serie B.

Signor Presidente, desidero intervenire su questo emendamento perché - secondo noi - tocca due temi particolarmente

con un massimo di due cittadini per ciascun genere, che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Perché sosteniamo questo emendamento? Lo sosteniamo per due motivi. Intanto, tocca un tema assolutamente fondamentale come quello della parità di genere, che non è di filosofia, per così dire - come credono molti, soprattutto in questo Governo - ma è banalmente di civiltà e di rispetto. Oggi il Parlamento italiano è fortemente maschile, è fortemente patriarcale ed è fortemente anche maschilista, in molti comportamenti che vediamo dichiarazioni che vengono rilasciate con grande leggerezza, da esponenti di questo centrodestra. Oltre a confermarlo i numeri, vi sono dei dati che dovrebbero indurvi a fare un ragionamento su questo. Sapete, andando avanti di questo ritmo, quando ci sarebbe parità di genere all'interno del Parlamento italiano? Quanti anni occorrerebbero per arrivare ad avere parità di genere nel Parlamento italiano? Andando avanti a questo ritmo, servirebbero centosessantadue anni. Io penso che il tema della parità di genere debba diventare una priorità per tutti

è oggettivamente, dal mio punto di vista, un fattore positivo, al di là delle legittime opinioni contrastanti. Credo, però, che, in assoluto, un Presidente del Consiglio donna sia un fattore assolutamente positivo.

Questo è il Governo che, pur avendo un Presidente del Consiglio donna, non si cura minimamente, ad esempio, del gap salariale all'interno del mondo del lavoro tra uomini in Italia le donne concludono gli studi prima degli uomini, e li concludono con un risultato migliore rispetto agli uomini; ma poi, nel mondo del lavoro, hanno molta più difficoltà rispetto agli uomini, ad esempio ad arrivare a raggiungere le posizioni apicali. Ed anche qualora ce la facciano, resta un *gap*, almeno del 30 per cento, nei salari rispetto agli uomini: questo è indecente. Questo Governo continua a dimostrare di non far nulla a tutela della parità di genere, quando, ad esempio, va a tassare i beni i beni per l'infanzia e i beni per la cura femminile, aumentando l'IVA, raddoppiandola, portandola dal 5 al 10 per cento. Quindi, la retorica del Presidente del Consiglio donna si ferma alla retorica, perché poi, nel merito, questo è un Governo che non fa nulla per la parità di genere. Questo è il primo punto dell'emendamento. Poi c'è una seconda parte, quella che restituisce i criteri per nominare i senatori a vita rispetto, tra gli altri, anche ai meriti artistici.

possiamo io, lei, può questo Parlamento arrogarsi il diritto di dire che figure - che hanno reso celebre l'Italia nel mondo per l'arte e la cultura - non hanno il diritto di diventare senatori a vita in Italia? Possiamo dire che il maestro Riccardo Muti non avrebbe titolo per diventare senatore a vita? Possiamo dire che il maestro Riccardo Muti potrebbe non portare un beneficio a quest'Aula? Ricordo che ieri il senatore Franceschini ha menzionato il maestro Claudio Abbado. Soprattutto l'Italia, queste figure, le deve valorizzare e certamente non cancellare, tra i requisiti per diventare senatore a vita, quello dei meriti artistici. Per chi, infatti, se lo fosse dimenticato - in questo Governo credo molti, sicuramente il Ministro della cultura - l'Italia è famosa nel mondo soprattutto per questi motivi; - come dice il maestro Muti - non è più famosa per essere il Paese della musica o dell'arte. Purtroppo, siamo famosi per essere il Paese della storia della musica e della storia dell'arte, perché ancora oggi godiamo dei benefici di cose accadute decenni e secoli fa.

ci dà sempre tanti spunti, così da farci superare la noia, andare avanti e trovare motivazioni per rispondere. Quella più facile è quando si riferisce alla Russia, chiedendo se quello è il modello a cui guardiamo. Ebbene,

in questa maniera. Ricordo - come abbiamo dichiarato - che noi lo facciamo perché siamo convinti che questa sia una battaglia per la difesa della nostra democrazia e della Costituzione. Torniamo a ribadire questi concetti, anche perché il segnale che deve passare fuori, nei confronti dell'opinione pubblica, è che noi ci batteremo fino in fondo per evitare questa che è una riforma sbagliata. La discussione è però anche utile per andare a rivedere e leggere il dibattito negli anni dell'immediato Dopoguerra, per comprendere come furono pensati i senatori a vita; fu non un capriccio, ma una discussione seria, un dibattito approfondito, nel corso del quale emersero anche visioni diverse. È vero che allora il Partito Comunista era contrario in nome del rispetto del principio di sovranità popolare, ma poi si trovò un compromesso. Lo stesso Togliatti chiese di trovare un compromesso rispetto alla proposta che veniva dall'allora Democrazia Cristiana e si ritrovarono su un punto: erano Costituenti che facevano sintesi, erano molto lontani, forse più lontani ancora di quanto si sia oggi, ma trovavano un terreno comune. Quello che stupisce invece del vostro atteggiamento è che continuate a rimanere arroccati sulle vostre posizioni e non fate un passo in avanti. *(Applausi)*. Questo è il punto fondamentale. Quando si parla di Costituzione bisogna trovare un terreno d'intesa comune.

lo hanno subito. È chiaro che, con un numero minore di senatori, anche il ragionamento sul numero dei senatori a vita

pensando alle riforme che ci sono state arrivare a quattro senatori e applicare la parità di genere, rende coerente l'assetto istituzionale rispetto alle battaglie che noi stiamo facendo, secondo dei princìpi che condividiamo. L'altro grande tema che viene meno anche rispetto a battaglie che avete fatto come centrodestra in passato è il ragionamento sulle sulle funzioni che i senatori a vita devono avere. Il dibattito in passato si è svolto sul fatto che potessero essere decisivi in alcuni passaggi parlamentari. Ebbene, voi non avete fatto nulla di tutto questo. Non vi siete chiesti come adeguare la figura dei senatori a vita alla nuova fase politica e istituzionale, alle nuove regole, alle revisioni costituzionali che nel frattempo si sono avvicendate. Avete fatto invece una scelta netta, eliminando figure come i senatori a vita, che invece sono delle personalità che arricchiscono il dibattito e contribuiscono in qualche modo a portare delle posizioni terze all'interno di quest'Aula. Rischiate quindi di sbagliare il bersaglio. In nome della sovranità popolare, private il Parlamento di personalità che possono arricchire il dibattito e permetterci di essere sempre più vicini alle istanze del popolo italiano. Per tali ragioni esprimeremo convintamente un voto

ma in realtà approfitto di questi minuti perché ho trovato, dal mio punto di vista, particolarmente stimolanti le riflessioni che ha fatto poco fa il Presidente della Commissione affari costituzionali cui in particolare, a quando ha fatto riferimento a un punto che, anche secondo me, avrebbe meritato un serio approfondimento e che davvero denota un elemento di differenza politica reale,

così ingenue da fare come hanno fatto l'ultima volta, cioè dividersi in quattro e in qualche modo favorire la vittoria delle destre. Insomma, ha motivato la natura stessa di questa riforma con una cosa, di cui abbiamo molto sentito parlare negli ultimi trent'anni: la cosiddetta democrazia dell'alternanza, che è una questione seria. Ora, io penso - ed è uno dei motivi di fondo, culturali, se posso dire, ancora prima che politici che politici - che il tema del cosiddetto bipolarismo rigido sia stato esattamente uno dei problemi politici con cui si è confrontata la nostra Repubblica negli ultimi trent'anni. Alla fine è stato questo il problema, è finita, sulle macerie di Tangentopoli, la prima Repubblica e da quando è nata la seconda Repubblica, fondata in qualche maniera sul sistema maggioritario e quindi sul bipolarismo. La tesi, all'epoca - devo dire - molto trasversale (c'era una sorta di pensiero unico su questo punto), che la semplificazione del bipolarismo rigido, alla fine, fosse di giovamento per la Repubblica italiana era molto popolare. Il *referendum* sul maggioritario del 1993 vide una altissima percentuale di favorevoli. È stata fondata una vera e propria ideologia attorno all'idea che il maggioritario e il bipolarismo dovessero produrre un quadro di semplificazione, costruito esattamente sulla tesi della democrazia dell'alternanza. Penso che noi saremmo dovuti partire esattamente da questo, da un bilancio di quello che è successo negli ultimi venticinque anni. Credo che il bipolarismo rigido - di cui ha parlato adesso il presidente Balboni - nel nostro Paese sia sostanzialmente fallito. Mi dovete spiegare perché avrebbe funzionato questo bipolarismo rigido: ha favorito la partecipazione popolare, tanto per dirne una, oppure ha accentuato l'astensionismo? Oggi una parte significativa del Paese non vota. vota. Ciò ha solo a che fare con le leggi elettorali? Ovviamente no: sarebbe sciocco e ingenuo credere che l'unica motivazione del distacco di larghissime fasce di popolazione rispetto alla vita pubblica abbia a che fare, semplicemente, con i meccanismi elettorali. Penso che sarebbe molto serio interrogarsi su questo, anche perché - ora sto finendo il tempo, ma il ragionamento è articolato e quindi lo continuerò nel prossimo intervento questo astensionismo sta assumendo sempre di più caratteristiche di censo. È come se tornassimo a centocinquant'anni fa, quando votavano solo i nobili, solo i ricchi. L'astensionismo cresce dove è più acuta la sofferenza sociale; i quartieri e i territori dove si vota di meno sono quelli più poveri, è là che si produce il distacco della popolazione dalla politica. fra poco, quando interverrò nuovamente sul successivo emendamento - che questo sia proprio un punto di differenza sostanziale, almeno per quanto riguarda me e il mio Gruppo. Noi non crediamo affatto che questa forzatura bipolare sarà un elemento di stabilità.

estremamente scivolosi. Vedo che anche oggi questa cautela non è presente tra noi. Mi riferisco in particolare - lo faccio con il massimo del garbo e della cortesia nei suoi confronti all'intervento del Presidente della mia Commissione, senatore Balboni, per giustificare il progetto governativo di oggi di eliminazione dei senatori a vita che sono stati introdotti dalla Costituzione del 1948, ha richiamato la posizione del Partito Comunista Italiano del 1946. Francamente, non non trovo che questo richiamo abbia un fondamento perché è davvero difficile giustificare questo intervento del 2024 con la posizione di un partito nel 1946. Siete un po' spericolati. *(Applausi)*. In termini di citazioni storiche fatte dal senatore Balboni, ho trovato molto più feconda e stimolante, per quanto mi riguarda, quella di Stanis Ruinas. Credo che in quest'Assemblea conosciamo solo io e il senatore Balboni il fondatore del "Pensiero nazionale". Quella era una citazione che, che, perlomeno, ci consentiva di approfondire un aspetto dell'opera di Togliatti nell'immediato Dopoguerra. In realtà, dobbiamo riconoscere dobbiamo riconoscere dei meriti al senatore Gasparri, che nel suo intervento ci ha spiegato, un po' tra le righe, ma chiaramente, il motivo vero per cui la destra in Italia ha messo all'ordine del giorno l'eliminazione dei senatori a vita. Il senatore Gasparri lo ha detto: il centrodestra vuole eliminare i senatori a vita

che non percepiamo come nostro, è addirittura venuto a votare la decadenza di Silvio Berlusconi. Questo è il livello della discussione che noi stiamo facendo *(Commenti)*, queste sono le ragioni profonde per le quali si pone il problema dell'eliminazione dei senatori a vita dal nostro ordinamento. *(Applausi)*. Vi siete posti a questo livello, che è del tutto legittimo, ma che trovo molto basso. Tirare in mezzo la sovranità popolare, lo sconvolgimento degli equilibri all'interno del Senato, la storia, la posizione del PCI nel 1946 e la posizione di un altro partito nel 1962 non ha alcun senso. La ragione vera è questa: qualche senatore della vostra parte l'ha detta e credo che dirla così chiaramente ci permette di fare un dibattito franco. I senatori a vita non li volete perché negli ultimi trent'anni avete percepito che il Presidente della Repubblica non ne ha nominato nessuno che poteva sembrarvi vostro. Quindi, è un'azione di rivalsa istituzionale. Questa è la ragione vera per cui volete eliminare i senatori a vita.

è l'occasione per ricordare loro che sono nell'Aula del Senato in un giorno importante: il giorno in cui ricorre, purtroppo, la morte di Giovanni Falcone, di Franca Morvillo e dei tre uomini della scorta, Montinaro, Dicillo e Schifani, che persero la vita per un drammatico attentato mafioso che colpiva loro per colpire la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra Costituzione, e per tentare di di sopravanzare la forza dello Stato. Noi li ricordiamo e nella loro memoria continuiamo in maniera inflessibile, stavolta tutti insieme, ad essere un baluardo contro l'eversione e la criminalità. Vi prego di osservare tutti insieme un minuto di silenzio nella loro memoria.

Sulla questione dei senatori a vita, noi facciamo una valutazione che è perfettamente lecita. Peraltro, anche i colleghi che ne difendono, nella prospettiva, la presenza, convengono che essi non dovrebbero votare per le votazioni di fiducia quantomeno, visto che in un Senato di 200 membri, con un numero variabile di senatori a vita, possono incidere. Non è un fatto teorico, perché tra il 2006 e il 2008 in quest'Aula (io allora ero alla Camera), la maggioranza del Governo Prodi si reggeva con un ricorso, a volte anche... Prego, a me piacciono le interruzioni.

Grazie Presidente. Stavo ricordando un fatto storico: ci fu una polemica, perché la senatrice Rita Levi Montalcini, una personalità eccelsa della Repubblica, giustamente premiata con quel riconoscimento, veniva spesso

dell'opposizione. Vi lamentate che non fa mai un intervento la maggioranza. Se quando lo fa interrompete, allora fanno bene a non parlare.

anzi, ho ascoltato l'intervento del senatore Franceschini che ha elencato i senatori a vita e ho citato - Presidente, lei non era in Aula - che lei per età ha detto di averne conosciuti numerosi. Io ne ho conosciuti alcuni, non quanti lei, ma abbastanza più di altri. Quindi, ho ricordato che Andreotti, quando ricordammo in Aula che compiva novant'anni, era seduto qui vicino, insomma si seccava che fosse ricordato il suo novantesimo anno, perché giustamente lo viveva come il tempo che trascorreva. Abbiamo avuto rispetto per il presidente Cossiga e per altri. Ho semplicemente constatato che, nell'elenco che ha letto il senatore Franceschini, non ho trovato alcune personalità culturali e politiche di un'area che ha governato per dieci anni il Paese. Era una lamentazione per una inclusione che io mi auguro. Se resteranno i senatori a vita, cosa che potrebbe accadere, mi auguro che si attinga a tutti i campi della scienza, dell'arte, della cultura del giornalismo. Credo sia un'opinione che si possa esprimere. Per quanto riguarda il senatore Renzo Piano, che potrebbe in questo momento venire in Aula e parlare, perché è senatore (giusto, no?), riscontrato la sua non intensa frequentazione dei lavori parlamentari, che non gli ha però impedito di venire in un'occasione significativa (era un suo diritto), in cui si votava la decadenza di Berlusconi. L'avrei voluto vedere quando si votavano provvedimenti per i poveri, per i terremotati, per le Forze di polizia. *(Applausi)*. Non mi pare però sia il caso di andare a esaminare le occasioni in cui ciascun senatore è stato presente o assente, perché tutti potremmo trovare elementi

Signor Presidente, le devo confessare che sono rimasta un po' interdetta per il fatto che, pur essendo iscritta prima di Gasparri, per un motivo che poi, forse, ci vorrà spiegare ha dato la parola prima

fatevi qualche domanda. *(Commenti. Applausi)*. Parto dalla fine, perché qui invece il presidente Balboni si rivolgeva in maniera indistinta verso i banchi del campo progressista, facendo riferimento alla Russia. La Russia è l'unico Paese che ha i senatori a vita, evidentemente facendo riferimento addirittura alla Russia sovietica. Ma l'esempio più vicino della Russia invece è Putin e io faccio presente al senatore Balboni e a tutti gli esimi colleghi e colleghe della destra che solo sei mesi fa il "lettone" di Putin è stato traslocato da Palazzo Grazioli di Berlusconi. Quindi eventualmente le contingenze e le vicinanze sono tutte vostre. Non solo. Tornando a rappresentanti culturali che potrebbero illustrare l'alto pensiero della destra italica, mi pare che sia ai vostri convegni e raduni che viene invitato l'ideologo russo Dugin, non ai nostri. *(Applausi)*. Quelli sono i vostri riferimenti culturali ed eventualmente dovreste cambiare la Costituzione per dire che i senatori a vita possono essere anche di altre nazionalità, segnatamente di nazionalità russa. Ma siccome ci è stato anche rinfacciato che noi, attraverso Vito Crimi, abbiamo depositato, non so quanti anni fa, un disegno di legge in cui abolivamo i senatori a vita, faccio presente innanzitutto che nella nostra riforma culturale quella che rivendichiamo con orgoglio, in cui abbiamo diminuito il numero dei parlamentari - evidentemente ci abbiamo pensato e abbiamo portato il numero dei senatori a vita ad un numero definito (cinque), che ci è sembrata una soluzione ragionevole e di compromesso per illustrare la Patria con chi si sia distinto. Ma, se parliamo di chi ha cambiato idea improvvisamente su tutto, io credo che Fratelli d'Italia non possa fare lezione proprio a nessuno, perché noi siamo qui a discutere di premierato, quando nel vostro programma c'è il presidenzialismo, che non è affatto la stessa cosa. Avete promesso di abolire le accise e mi pare che le accise non si siano mosse: il prezzo della benzina e del *diesel* è altissimo. *(Commenti)*. Avete promesso l'abolizione dell'IVA l'abolizione dell'IVA sui prodotti per l'igiene femminile e per l'infanzia e invece l'avete rialzata. *(Applausi)*. Ma, soprattutto, Giorgia Meloni nel 2014 ha depositato un disegno di legge, con tanto di conferenza stampa e video, per

ovviamente molto interessanti - del presidente della 1a Commissione Balboni e in particolare, come ha fatto già il collega De Cristofaro, per questo suo riferimento alla democrazia dell'alternanza. anch'io sposo l'idea che la democrazia dell'alternanza sia una finalità da condividere, per così dire, ma soltanto se per democrazia dell'alternanza pensiamo a una democrazia nella quale, al contrario di quello che è successo in Italia per i primi cinquant'anni della Repubblica, c'è qualcuno che governa sempre e qualcuno che sta sempre all'opposizione, e ciò perché questo non è un modo sano di gestire una Repubblica democratica: infatti che, se ogni tanto non c'è qualcuno che dà aria alle stanze e apre gli armadi, evidentemente possono crearsi situazioni distorsive. Va benissimo quindi pensare a una democrazia in cui si alternano destra e sinistra al Governo; fatto che la democrazia dell'alternanza sia sinonimo di un bipolarismo spinto al bipartitismo nutro però qualche dubbio. Devo dire la verità: la verità: in teoria non ho antipatia per le democrazie che ruotano intorno a sistemi bipartitici; penso che abbiano il loro senso e siano spesso tra le più nobili esperienze di democrazia che conosciamo

bipolare, perché non mi sembra che abbiano funzionato benissimo e le ragioni potrebbero essere molteplici (forse ce n'è una anche di tipo culturale). Io, per esempio, mi stupisco moltissimo ogniqualvolta in campagna elettorale mi trovo in Comuni con meno di 15.000 abitanti, dove c'è una legge maggioritaria secca, diciamo quasi britannica, perché mi viene da pensare che un meccanismo di questo genere incoraggi la formazione di due liste concorrenti, mentre capita tantissimo nei Comuni, anche piccoli, che, pur in presenza di una legge siffatta, si presentino quattro liste diverse, cosicché diventa sindaco chi ha preso il 26

ci sono momenti nei quali le divisioni, anche all'interno delle stesse coalizioni, sono sui valori o su questioni legate all'estrema complessità del nostro tempo.

omogenei degli ultimi tempi: pur essendo la Lega e il Movimento 5 Stelle appartenenti a due schieramenti diversi, certe pulsioni antisistema - e un certo spirito rivoluzionario, per così tutto quello che si faceva prima non andava bene e bisognava cambiarlo - sono state un cemento più forte anche delle collocazioni politiche nelle quali i due partiti si trovavano. In conclusione allora, Balboni - fate attenzione a pensare che un accrocchio meccanicistico possa costringere forze politiche così diverse a diventare due poli o addirittura due partiti, perché in realtà le cose non sono così semplici.

certamente non solo per il rispetto enorme, il ricordo e l'omaggio che sento che il Paese intero debba a Rita Levi Montalcini. La *verve* che ho messo nella questione, infatti, è legata anche al fatto che che il Governo che è stato citato, guidato dal presidente Prodi, è caduto anche grazie a una compravendita, proprio di senatori. Ed io ritengo che ci siano poche cose che feriscono la democrazia quanto comprare senatori.

e che ovviamente veniva tenuto aperto. Adesso vi interessa tanto la stabilità, ma, evidentemente, la stabilità del Governo non era un bene quando governava Prodi, perché in quel periodo, appunto,

la democrazia si deve accompagnare alla libertà; dalle parole con le quali qui oggi la maggioranza chiede l'abolizione della figura del senatore a vita emerge invece un'insofferenza nei confronti della libertà, per cui i senatori a vita vanno bene solo se fanno quello che vuole la maggioranza.

in ascolto delle considerazioni fatte dal presidente Balboni, poi riprese anche dal senatore Scalfarotto. Secondo me, esse sono esattamente al centro della riflessione che facciamo o che dovremmo fare e che denotano questo grande punto di differenza. Non credo che questa democrazia dell'alternanza di cui voi parlate possa vivere in una fase storica come questa. Mi spiego meglio: non credo che una fase storica come questa, segnata dai fenomeni di cui parlavo prima, innanzitutto l'astensionismo dilagante, ferita gigantesca per la democrazia di questo Paese, possa essere risolta dalla scorciatoia dell'elezione diretta. Questo è il vero punto di differenza che probabilmente c'è tra di noi. Su questo, vi invito a fare una riflessione su quello che accade fuori dai confini nazionali. Il senatore Parrini ieri ha spiegato, secondo me molto bene, perché sistemi e forme di Governo esistenti in altri Paesi, puramente presidenzialisti, che pure non ci piacciono, hanno però una serie di pesi e di contrappesi che in qualche modo le rendono meno permeabili a possibili elementi di torsione. Il senatore ha fatto il caso di quei sistemi puramente presidenzialisti in cui alla forte concentrazione di potere che esiste, per esempio, in quel caso specifico nelle mani del Presidente degli Stati Uniti d'America - corrisponde un altrettanto forte concentrazione di poteri che c'è nei confronti del nei confronti del Congresso americano. È il tipico esempio, dice il senatore Parrini e secondo me dice bene, di un sistema presidenzialista che però in qualche modo prevede un elemento di pesi e di contrappesi e un equilibrio di potere che rendono quel sistema meno permeabile a possibili elementi di ritorsione. La riflessione che avremmo dovuto fare noi

finanche in un sistema puramente presidenzialista, con i pesi e i contrappesi come quello americano, segnalano degli elementi problematici, cosa potrebbe succedere in un sistema ancora più squilibrato come quello che volete presentare?

un sistema rigidamente di pesi e di contrappesi? Che cosa sta accadendo praticamente in quel Paese? Sta accadendo che la fluidità della democrazia contemporanea, anche lì, sta determinando elementi di lacerazione che l'elezione diretta amplifica; non vi sono invece elementi di lacerazione che l'elezione diretta riduce. Pensate ai due elettorati: all'elettorato che voterà da qui a pochi mesi il candidato del Partito Repubblicano e all'elettorato che voterà il candidato del Partito Democratico. La stragrande maggioranza degli elettori che voteranno il candidato democratico ritengono che il candidato dei conservatori andrebbe arrestato e messo fuorilegge. La stragrande maggioranza degli elettori che voteranno La stragrande maggioranza degli elettori che voteranno il partito repubblicano ritengono che il candidato democratico sostanzialmente dovrebbe essere messo da parte perché poco capace di intendere e di volere. Io non sto dando giudizi di merito sull'uno o sull'altro: sto semplicemente dicendo qual è la narrazione che c'è in quel Paese tra i due differenti blocchi. Questa cosa vuol dire che anche una democrazia come quella, quando subentrano elementi di lacerazione così forti, inevitabilmente si espone a possibili torsioni poco democratiche. Questo è il punto su cui state riflettendo poco. *(Applausi)*. Non voglio dire che la destra italiana porta con sé il germe della torsione antidemocratica. Non voglio dire questo. Voglio dire che si sottovaluta: ... ho finito, ma è un punto importante del ragionamento...

pertanto lei non abbia avuto modo di ascoltare tutti gli interventi. In uno di questi, proprio oggi nella ricorrenza che ha messo bene in evidenza lei, la strage di Capaci,

altro rappresentante di partito, dicendo che potremmo anche proporre il generale Mario Mori come senatore a vita. Senza nulla togliere, al di là del fatto che già nel 2021 il

perché noi rispettiamo le prerogative dei poteri dello Stato: siamo anche noi garantisti, perché non c'è una primazia tra chi lo è di più e chi lo è di meno. Siamo per il rispetto delle regole e oggi ci sembra inopportuno che in quest'Aula si facciano queste provocazioni, anche perché nelle ultime settimane abbiamo visto che il generale Mori è indagato dalla

Segre dare una lezione a tanti di noi, almeno a me sicuramente. Con il suo intervento, con la sua memoria, con il suo vissuto, ha fatto ancora una volta capire l'importanza di di come è stata costruita la nostra bella Carta costituzionale e di come, invece, questo Governo, in maniera improvvida, con i suoi Ministri e con questa maggioranza, continua a giocare con

non come battutine spicciole, ma a microfono attivo, perché noi siamo qui anche per argomentare e controbattere. Noi pertanto siamo favorevoli al mantenimento della prerogativa del Presidente della Repubblica per la nomina di altissime personalità

Signor Presidente, visto che si parlava del generale Mori, mi piacerebbe sapere come mai il dottor Tescaroli non sia ancora andato a Prato, dopo che è stato nominato da mesi: ma questa è un'altra questione di cui parleremo col ministro Nordio. Vorrei soltanto completare il ragionamento che facevo prima sulla democrazia dell'alternanza, o meglio sul bipartitismo, che, secondo il senatore Balboni, questa riforma rafforzerebbe: un bipolarismo spinto che meccanicamente si introdurrebbe. Prima dicevo che forse c'è anche una componente culturale tra noi italiani, che siamo abituati a dividerci anche quando siamo in pochissimi.

i sistemi bipartitici o tendenzialmente tali si sono giovati storicamente anche di una tendenza che portava questi grandi agglomerati ideali a tendere verso il centro. Che cosa accadeva? Nel Partito Democratico americano un democratico del Maine era sicuramente più a sinistra di un democratico dell'Alabama e il democratico dell'Alabama spesso era più a destra del repubblicano del Maine. Accadeva infatti che dentro questi grandi corpi elettivi erano rappresentate posizioni diversissime, ma il sistema politico tendeva a trovare dei punti di sintesi che fatalmente portavano i partiti a spostarsi verso il centro. Vi

sono fortissime. Pochi minuti fa Nikki Haley ha detto che voterà per Trump, quindi la speranza di avere una anti-Trump nel Partito repubblicano è sparita. Nel Partito Democratico Democratico americano, personaggi come Alexandria Ocasio-Cortez o come lo stesso Bernie Sanders, che hanno avuto un grande impatto e una grandissima popolarità, hanno posizioni - e grazie a tali posizioni hanno ottenuto quella popolarità - molto polarizzate. Vogliamo guardare alla Gran Bretagna? Guardate che la resa dei conti tra Starmer e Corbyn avviene non su un tema economico o su un tema di secondaria importanza; Corbyn viene accusato di antisemitismo,

quando il Regno Unito stava nell'Unione europea e utilizzavano il proporzionale soltanto per le elezioni europee (l'unico caso in cui dovevano usarlo per forza), la destra di Nigel Farage andava sempre fortissima. Vogliamo guardare che cosa sta succedendo in Germania con AfD, che in molti Länder supera il 20 per cento? Dobbiamo renderci conto che quella tendenza - secondo me virtuosa, ma forse secondo il collega De Cristofaro meno

Ci sarebbero forze politiche da questa parte dell'Emiciclo e da quell'altra parte che voterebbero insieme, contrariamente alla loro collocazione. Allora attenzione, perché credo

vita. State sottraendo una prerogativa al Capo dello Stato e state portando un attacco al Presidente e alle sue prerogative. Che cosa farà il Presidente della Repubblica dopo che gli avrete tolto questa prerogativa? Cosa potrà fare? Potrà nominare dei cavalieri del lavoro, ma, oltre a ciò, non potrà più incidere.

Ebbene, su 146 Paesi, nessun Paese del mondo, compresa l'Italia, ha mai raggiunto la piena parità di genere e ci vorrà un secolo per raggiungerla.

nominare cittadine e cittadini, alternando maschi e femmine. Questa è una prerogativa che noi vogliamo dare al Capo dello Stato, per consentire una vera parità di genere, che è indicata come priorità dall'Agenda 2030 in tutto il mondo. *(Applausi)*. Il World Economic Forum ha detto che una delle priorità, che deve incidere anche nelle istituzioni politiche come cambiamento culturale, sta nel portare a una parità di genere. Ripeto che voi volete sottrarre la prerogativa al Capo dello Stato di introdurre la possibilità di una parità di genere tra i

Forse questa maggioranza non sa che l'Italia ha perso ben 13 posizioni, scivolando, tra i 146 Paesi del mondo, alla settantanovesima posizione.

è l'assoluta mancanza di volontà di provare a fare un bilancio, intellettualmente onesto, di quello che è successo in Italia negli ultimi venticinque anni e di dove sono annidate le cause dell'allontanamento sempre più clamoroso di milioni di persone rispetto alla politica, ai partiti e alle elezioni, visto che l'astensionismo cresce in maniera gigantesca. Per inciso, cresce in maniera gigantesca anche in caso di elezione diretta,

vive la maggioranza di elettori che non si reca alle urne e scoprirete che si trova dove è più forte la sofferenza sociale e dove ci sono più povertà, maggiore evasione scolastica e più povertà educativa. Questo sta succedendo in Italia:

erano solo coloro che avevano i soldi e una precisa connotazione di censo. Questa è la fotografia della realtà: non è una ricostruzione di parte, ma è un dato oggettivo che si apprende semplicemente guardando i dati elettorali. la domanda è: rispetto a questa crisi così evidente e rispetto al fatto che qualche decennio fa i cittadini iscritti iscritti ai partiti politici in Italia erano circa 15 milioni e oggi tutti insieme non arrivano a un milione; dinanzi alla crisi totale dei corpi intermedi, dei luoghi plurali, delle "casematte" di tutto quello che nel corso del '900 ha contribuito a costruire la democrazia italiana, davvero si può pensare che la scorciatoia dell'elezione diretta risolva questo problema e invece non lo accentui? Davvero si può non comprendere come, in una società così liquida, così destrutturata, così lacerata, quella scorciatoia rischia di portare esattamente alla condizione di cui ho parlato prima, quella degli Stati Uniti d'America, dove ci sono due elettorati che pensano il peggio possibile l'uno dell'altro? Credo che queste siano grandi domande aperte, sulle quali avremmo dovuto interrogarci, perché sono le domande di fondo che attraversano oggi la qualità della democrazia di questo Paese. Come si fa a non vedere che questi sono i temi di cui si discute in tutta Europa, anche in quei Paesi dove esiste il presidenzialismo e dove, non a caso, aumentano le voci di quelli che stanno facendo suonare i campanelli d'allarme, esattamente perché stanno comprendendo - ho finito gli elementi di esposizione alle possibili torsioni autoritarie aumentano? Questa è la domanda di fondo, ma purtroppo a questa riflessione non si dà - almeno a mio avviso - un'adeguata risposta. Si cerca soltanto una scorciatoia molto demagogica.

necessariamente la soluzione ideale. Lo dico perché il senatore Balboni, tra le altre cose, Presidente, faceva notare una unità di questa maggioranza a fronte della divisione dell'opposizione e diceva: dovreste quasi ringraziarci, perché, grazie a questo accrocco ingegneristico, sarete costretti a mettervi insieme. Io invece penso che le cose anche qui non siano così semplici. Il collega De Cristofaro faceva riferimento alla crisi della politica. Secondo me, la crisi della politica sta anche nel fatto che, se non è bene che le possibili coalizioni siano frammentate, non è neanche tanto bene quando ci sono delle coalizioni che stanno insieme senza un cemento programmatico sufficientemente forte. La maggioranza così coesa che descrive il presidente Balboni forse la vedono i colleghi della maggioranza in quest'Aula; ma il fatto che non esista è davanti agli occhi del Paese. Per esempio, sulla leva obbligatoria qual è la posizione della maggioranza? Non ho ben capito se siete d'accordo o no. Sul redditometro mi piacerebbe sapere se le indicazioni del vice ministro Leo siano condivise da questa maggioranza così così coesa. Sul sostegno militare all'Ucraina, precisamente la posizione della maggioranza io ancora tanto bene non ho capito quale sia. E c'è tutta una serie di argomenti, sulla quale potremmo intrattenerci, che ci fa vedere che l'azione del Governo è in difficoltà. Me ne viene un altro:

dei parlamentari, noi siamo abbastanza soggetti ai cicli vitali del collega Lotito, a seconda di quando è più pimpante e di quando lo è un pochino meno, perché i numeri in Commissione bilancio, diciamo così, sono piuttosto ballerini. Per non parlare delle feste di compleanno di Damiani,

cada. La cosa che non va bene è quindi pensare che, dato che abbiamo sistemi che costringono le coalizioni a stare insieme anche contro i loro programmi, questo possa riqualificare la politica e fare in modo che le nostre lise istituzioni possano recuperare uno smalto che non hanno più. Ribadisco allora di ritenere che questa riflessione dovremmo fare e dovremmo ragionare sulla crisi della politica più in profondità. profondità. E lo dico da parte di un Gruppo convintissimo che sia fondamentale non perdere altro tempo e fare le riforme costituzionali, che l'assetto istituzionale del Paese sia in sofferenza,

che ha presieduto un ramo del Parlamento, per noi, dal nostro punto di vista, doveva essere la grande occasione per un'ampia riflessione che andasse alle radici del problema. C'è invece la sensazione che questa sia la classica riforma sintomatica, un po' come l'aspirina o la tachipirina: come quella roba che magari prova ad abbassare la febbre, ma non cerca la cura dell'infezione e la rimozione delle cause della malattia. Probabilmente quindi, come quando prendiamo la tachipirina, ci ritroveremo dopo poco punto e daccapo. il Partito Democratico ha elaborato questo emendamento, che ho già illustrato ieri, con l'obiettivo di preservare le prerogative del Presidente della Repubblica, assicurare la partecipazione di figure autorevolissime della nostra Nazione alla vita istituzionale ed esplicitare l'importanza dell'accesso delle donne alla nomina di senatrici a vita, a fronte di un passato che - come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto - come in tutti gli ambiti in cui sia riconosciuto un qualche grado di autorità, le ha viste sempre in netta minoranza rispetto alla parte maschile. signor Presidente, all'interno del nostro corpo degli emendamenti, senza dubbio di portata notevole, nella prospettiva - speriamo non del tutto vana - di arginare l'azione scellerata di questo Governo: essa è volta a cambiare l'assetto strutturale della nostra democrazia rappresentativa

si pone in aperto contrasto con le rassicurazioni, più volte ribadite dalla maggioranza, sul mantenimento delle prerogative del Capo dello Stato. Non solo propone di abolire la carica di senatore a vita, ma sottopone anche a vincoli stringenti la nomina del Presidente della Repubblica e la possibilità di scioglimento delle Camere: in favore di un assetto formale della Repubblica, con il quale illudete elettrici ed elettori di restituire loro un fantomatico maggiore potere. Come ho ribadito qualche giorno fa in quest'Aula - e non sono stata la sola - tutto ciò costituisce solo un maldestro tentativo di gettare fumo negli occhi ai cittadini e alle cittadine, perché non avranno alcun potere in più; semmai, il contrario: li costringerete a un'unica votazione maggioritaria ogni cinque anni, cioè a decidere sulle proposte dei vertici del sistema politico senza avere, successivamente, modo di manifestare il proprio giudizio e la volontà popolare. Il vostro disappunto è destinato a continuare, colleghi e colleghe della maggioranza, perché non smetteremo mai di ricordarvi che la Carta costituzionale è stata pensata, ideata e iscritta per tutelare il nostro Stato da quei ritorni di uomini - e donne - soli al potere su cui tanto vi piace fantasticare. E poco importa se quelle donne, quando arrivano al potere, dimenticando convenientemente di aver giovato dei sacrifici e delle lotte di chi li ha precedute nel costruire la nostra democrazia, proprio come le ventuno Costituenti, su un totale di 556 deputati eletti all'Assemblea:

Noi non dimentichiamo, invece, quel sacrificio e quelle lotte e continueremo ad opporci ai tentativi di chi vorrebbe renderli vani. Signor Presidente, proprio perché nel nostro articolo, che prevede quali sono i requisiti

Qui non ci sono vittime e carnefici. In quest'Aula si fa altro. Allora, io forse faccio, non un'altra provocazione, ma un'altra proposta. Se fossero stati vivi i nostri Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo,

dare continuità e riconoscibilità a chi ci sta seguendo qui in Aula e ai cittadini, non me ne voglia il collega senatore De Cristofaro, ma il voto di Azione è in senso difforme è in senso di astensione. Come lei sa, signor Presidente, noi siamo molto contrari alla soppressione di una delle prerogative del Presidente della Repubblica, sulla nomina dei senatori a vita. Dall'altra parte, noi riteniamo che, pur essendo legittimo l'approccio ostruzionistico fatto dalle opposizioni, questi emendamenti non siano quello che ci servono. il fatto di non aver apportato una modifica sull'alternanza di genere, tra i cittadini e le cittadine, non ha in alcun modo impedito ai Presidenti della Repubblica di nominare senatrici a vita come Liliana Segre, come Elena Cattaneo, come Rita Levi Montalcini e tutte quelle che abbiamo citato. è un messaggio che - secondo me - è importante anche per tutte le cittadine italiane che ci seguono. Non è tanto una modifica di una parola nella Costituzione, ma è la capacità di contraddistinguersi in maniera da illustrare la Patria ai sensi della Costituzione, il criterio che deve consentire al Presidente della Repubblica di nominare senatrici a vita che possono illustrare la nostra Patria. Ecco perché, signor pur rimarcando la contrarietà di Azione a questa posizione della maggioranza, alla quale noi siamo assolutamente contrari, pensiamo che già oggi la nostra Costituzione garantisca le elezioni delle senatrici a vita: quindi voteremo in astensione rispetto a questo emendamento.

siano parole al vento, dal momento che questo Governo sta narcisisticamente guardando se stesso allo specchio e non vuole accettare suggerimenti, neppure dai parlamentari della maggioranza. considerate questa come la madre di tutte le riforme. Io non so se ci rendiamo davvero conto di cosa significa "madre di tutte le riforme". È come dire che il problema italiano

e condizioni di sviluppo nelle aree dove ci sono carenze infrastrutturali. Avete bocciato tutti gli emendamenti che avevamo presentato nella riforma dell'autonomia differenziata per fare in modo che tutte le Regioni avessero le stesse possibilità di sviluppo. No. Qual è il problema dell'Italia? Dove incide questa madre di tutte le riforme? Il problema dell'Italia è la Costituzione, è l'equilibrio costituzionale, è una Costituzione democratica, che non consente l'autoritarismo. Volete rompere quegli equilibri. La madre di tutte le riforme è il ritorno a figure autoritarie.

provate a sentire che cosa ci dice l'Europa. Presidente, io non riesco a nascondere l'imbarazzo che ho provato a un incontro interparlamentare a Bruxelles in cui si parlava dello Stato di diritto, quando uno dei relatori, parlando dell'Italia, ha detto che nel nostro Paese si utilizzano troppi decreti-legge, che c'è un abuso della decretazione di urgenza. Dobbiamo farcelo dire dall'Europa? Non siamo in grado da soli di rimediare a questa incongruenza democratica? Voi invece la stabilizzate. Avete respinto già in Commissione un emendamento della senatrice Maiorino che proponeva un piccolo rimedio, cercando di dare omogeneità ai decreti-legge. Ce lo ha detto l'Europa. No: voi non ascoltate nessuno, non ascoltate i vostri parlamentari a cui non date possibilità di emendare, non ascoltate le opposizioni e non ascoltate neppure l'Europa. Ancora, la democrazia - come ci dice l'Europa e anche qui faccio riferimento a quello che hanno detto in Europa durante un incontro interparlamentare - è fatta di democrazia rappresentativa (di qui l'importanza del Parlamento), ed è fatta anche di democrazia partecipativa. In uno dei *dossier* europei si dice che l'Italia non è così vitale nel dare ascolto alle petizioni, non c'è una vera e propria democrazia partecipativa. Che cosa state facendo al riguardo? Niente: voi fate una riforma dove i cittadini saranno sempre più esclusi, perché saranno esclusi dalla vita politica i loro rappresentanti, che non conteranno più nulla, e non c'è nulla che possa andare a rafforzare il potere dei cittadini e i loro strumenti di partecipazione democratica. Presidente

capisco, ma a me sembra che questa riforma più che altro sia bipolare. Questo Governo sta facendo una riforma che fa seguito a una riforma diametralmente opposta; da un lato, volete togliere potere a Roma ladrona, la Lega vuole decentrare il potere e, dall'altro, volete fare una concentrazione del potere non nelle istituzioni democratiche, ma in una sola persona che avrà il potere di mandare a casa il Parlamento senza alcun potere discrezionale. Qui non è discrezionalità. È arbitrio perché, se voi non mettete nero su bianco quando questo potere può essere esercitato *(Applausi)*, significa che il Presidente del Consiglio può decidere di dimettersi da un giorno all'altro e mandare tutti a casa senza alcuna ragione. senatore Malan che il Presidente della Repubblica nel nominare senatori a vita per gli altissimi meriti - come recita la nostra Costituzione - debba attenersi all'alternanza di genere. Si parla di limitare i poteri del Presidente della Repubblica e questa è una limitazione fortissima su un aspetto estremamente delicato. se il presidente Napolitano avesse nominato la senatrice Cattaneo senatrice a vita come ultima del suo mandato, invece forse era la penultima, il presidente Mattarella non avrebbe potuto nominare Liliana Segre senatrice a vita per ragioni di alternanza, che lo stesso Napolitano, non ancora senatore a vita, non ancora Presidente della Repubblica, nel 2005 non avrebbe potuto essere nominato senatore a vita perché prima era stato nominato Mario Luzi. Ecco, si dice di voler limitare i poteri del Presidente della Repubblica, ma qui andiamo anche oltre. Poi ho visto che più in là ci sono anche delle proposte, degli emendamenti autorevolmente firmati, in cui si afferma che devono avere almeno settant'anni, probabilmente per garantire l'idea di un ricambio, di un ricambio, contando sul fatto che la vita umana ha un limite. Immagino che sia quella la ragione, perché ci sono sicuramente delle persone validissime con altissimi meriti, alcune delle quali

visto che c'è molto perbenismo da parte della opposizione, pregherei che ci sia anche un pochino di coerenza; altrimenti, se presentate gli emendamenti solo per guadagnare tempo, questo è un altro conto, è un diritto, ma è anche nostro diritto far notare le gravi incongruenze che ci sono.

il Parlamento analizzasse cosa è avvenuto in tutti questi anni e perché, non solo nella politica ma anche nella società, c'è una crisi della rappresentanza.

ma io credo che la democrazia sia prima di tutto rappresentanza, e quindi richiede che tutti i soggetti siano rappresentati in modo proporzionale al loro peso. Ritengo che la democrazia sia, invece, partecipazione,

tra i lavoratori e le lavoratrici. Tuttavia, se qualcuno pensa che si possano imporre le scelte, in questo caso viene meno la democrazia. Questo problema lo abbiamo noi, ma lo hanno anche le forze sociali. è vero che c'è una crisi della rappresentanza nel mondo sia sindacale che delle imprese? È chiaro che c'è una parcellizzazione, una frantumazione, per cui facciamo fatica a

dovremmo discutere con molta più passionalità, determinazione, ma nello stesso tempo avere capacità di ascolto, per favorire il livello partecipativo. La partecipazione è democrazia, è un anticorpo contro l'autoritarismo, è la cosa migliore per

di fare un passo indietro rispetto a questa discussione che non ci porterà alla soluzione. Si pensa che l'uomo o la donna forte risolva il problema della complessità della società? Ho citato prima Ho citato prima operai e impiegati, ma vogliamo parlare dei giovani? Quanti giovani ci sono in questo Parlamento? Quanti immigrati ci sono in questo Parlamento? Eppure la nostra società ne è piena. In sostanza, noi rappresentiamo realmente la composizione della società?

Spero che i giovani si ribellino a questa impostazione.

una narrazione che ci convince estremamente poco ed è anche un'opportunità per porvi alcune domande, nella speranza che possano suscitare nei vostri animi un dubbio e, chissà, forse un ravvedimento. Il racconto che voi fate al Paese è sostanzialmente questo: "Noi siamo i cantori, i bardi, i difensori, i fautori della sovranità popolare per questo proponiamo che il Presidente del Consiglio sia eletto direttamente dal popolo", anche se non lo fa nessun Paese nel mondo in cui ci sia, insieme al Presidente del Consiglio, un Presidente della Repubblica. Per questo sostanzialmente dite: «Vogliamo un Senato esclusivamente elettivo. Quindi è in nome della difesa della sovranità popolare che noi proponiamo l'espulsione dal Senato di chiunque non abbia avuto l'unzione di una elezione popolare e quindi la giustificazione, il bagno di legittimità, che la sovranità popolare produce». È una propaganda ingannevole, ovviamente, ma ha il suo fascino. Credo che però sia molto facile dimostrare che tutte le scelte che avete fatto all'interno di questa operazione di riforma costituzionale vanno esattamente contro la difesa della sovranità popolare, ed è in questo senso che spero che le parole che sto per dire possano suscitare un ravvedimento nella maggioranza. Faccio il primo esempio: sono mesi che il Governo si rifiuta di rispondere a una semplice domanda che il Partito

che c'è in tutte le democrazie in cui si elegge direttamente una carica monocratica nazionale? Vi siete rifiutati di mettere il 50 per cento in Costituzione perché avete in mente di rendere possibile l'elezione a minoranza di un *Premier* con molto potere, perché perché questo significherebbe una soglia inferiore. La domanda che vi faccio è la seguente: ma un *Premier* che venisse eletto direttamente a Palazzo Chigi con il 41 per cento dei voti, e che avrebbe contro quindi il 59 per cento degli italiani, è un omaggio alla sovranità popolare o o un modo di calpestare la sovranità popolare? Vi rendete conto della gravità dell'operazione che avete in mente? Lo sanno anche i bambini che avete in mente il 40 per cento e che non accetterete mai la soglia della metà più uno per legittimare il conferimento di così tanto potere alla carica che sta al vertice del potere esecutivo. Un *Premier* che va a Palazzo Chigi con la maggioranza degli italiani contro è un modo di violentare la sovranità popolare, non un modo di inchinarsi alla sovranità popolare. Vi è una seconda questione che dimostra la vostra malafede politica: non avete voluto prendere in considerazione il nostro invito, ripetuto più volte, non dico ad esaminare insieme, ma ad affiancare alla discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935 la presentazione di un disegno di legge di riforma della legge elettorale per eleggere i parlamentari. A questo punto, siccome i nostri appelli cadono nel vuoto da mesi, ci siamo fatti delle domande: come mai si rifiutano di mettere nero su bianco che tipo di riforma elettorale vogliono? Ne abbiamo avuta una testimonianza nel dibattito che si è svolto fin qui: perché tra di voi non siete d'accordo. Il senatore Balboni ha proposto le preferenze; il senatore Malan vuole il Mattarellum, ma non si è accorto che, per come è scritto l'articolo 5, il Mattarellum non si può applicare (glielo ricordo, prenda nota); gli altri partiti non dicono niente perché, come sappiamo, non vogliono rinunciare alle liste bloccate, nemmeno sotto tortura. Anche questa oscurità, nella quale lasciate la modalità con cui si eleggeranno i parlamentari, quindi l'Assemblea che rappresenta tutto il popolo, è un modo non di rendere omaggio, ma di violentare la sovranità popolare, e fa capire che siete in malafede. La terza questione è l'elezione a strascico del Parlamento. Come si può pensare che sia una maniera di...

cercando di argomentare sempre meglio il ragionamento, in quanto molto spesso i tempi ci costringono ad abbreviare e a sintetizzare. Ho detto prima che la democrazia è un fatto complesso.

sostituite e sono nati i consigli di fabbrica, che erano diversi: le commissioni interne erano liste delle associazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, mentre i consigli di fabbrica erano eletti dai lavoratori su scheda bianca. Vi garantisco che fare la sintesi da quel punto di vista era più complesso, ma era più veritiero.

i soggetti, le persone che sempre meno partecipano alla vita politica. Sono le persone che vivono una situazione di abbandono scolastico e di difficoltà ad arrivare a fine mese, che vivono nelle case popolari, e che comunque percepiscono una cosa: che tanto la politica per loro non cambia nulla. Partecipando o no, la loro condizione non trova una modificazione e per questo delegano.

in modo antidemocratico. Io francamente penso che la democrazia sia un'alternanza e che sia giusto avere delle opinioni diverse. Credo che la politica è passione, è parte,

durante la discussione svolta in Commissione abbiamo cercato di far emergere la contraddizione tra ciò che cercate di raccontare ai cittadini e ciò che la riforma è. Lo ha ricordato adesso, peraltro in maniera molto efficace, anche il senatore Parrini. La narrazione di una maggiore attenzione alla sovranità popolare e del conferimento ai cittadini di un maggiore potere politico si scontra in maniera evidente con il contenuto della riforma, che finisce per concentrare tutto il potere in una sola figura e, soprattutto, esaurire la partecipazione politica e democratica nel momento delle elezioni.

come intendete risolvere alcune contraddizioni e aporie presenti nel disegno di legge. Devo dire che nel corso del dibattito di questa mattina, forse qualche informazione in più l'abbiamo potuta raccogliere perché

tempo. Se diamo credito alle parole che abbiamo ascoltato, io sono rimasto molto colpito dall'intervento fatto fatto dal senatore Gasparri per spiegare le ragioni della contrarietà al permanere delle prerogative, in capo al Presidente della Repubblica, di nominare fino a cinque senatori a vita. Mi ha colpito non tanto l'argomento (che è

un senatore di tale esperienza possa intervenire in quest'Aula e dire «se i senatori a vita resteranno, cosa che potrebbe accadere», così, con leggerezza. Qui si apre uno dei tanti profili che questo dibattito forse alla fine, stupendoci, potrebbe rivelare, cioè che sta maturando dentro la maggioranza la consapevolezza della necessità di rivedere parte significativa della riforma. sarebbe bene che, se questa consapevolezza sta crescendo, noi non fossimo costretti a rimanere qui a discutere di un testo che la stessa maggioranza già considera in parte superato. Questa considerazione, Presidente, vale anche per l'altra questione che vi siete rifiutati di trattare, quella della legge elettorale. Anche su questo punto, come ricordava prima il senatore Parrini, abbiamo chiesto più e più volte di conoscere quali sono le caratteristiche di fondo della legge elettorale che avete in mente e che dovrà essere coerente con il nuovo testo. Questa mattina abbiamo sentito, per bocca del relatore, dire che comunque la nuova legge elettorale non prevedrà l'attribuzione di un premio di maggioranza superiore al 15 È un'affermazione impegnativa, Presidente, detta dal relatore, che probabilmente è a conoscenza di una maturazione del confronto politico all'interno della maggioranza che quest'Aula purtroppo non ha potuto condividere. Se il relatore ci dice che la nuova legge elettorale non prevedrà comunque un premio superiore al 15 per cento, noi dobbiamo credere a questa affermazione. Ma allora, se è così, io chiedo ci si potrebbe anche dire, Presidente e relatore, come è... Lo dirà nel prossimo emendamento, grazie.

mi avrebbe fatto molto piacere occupare questa Assemblea per parlare dello sciame sismico che sta colpendo la zona dei Campi Flegrei. *(Applausi)*. Avrei colto l'occasione anche di poter in qualche modo interagire con il ministro Musumeci, visto e considerato che in questo momento mio figlio un istituto scolastico proprio in quella zona. Quindi chiaramente capisce bene che, secondo me, ci dovremmo occupare di questi argomenti, oltre al fatto che purtroppo a Napoli, proprio ieri, siamo stati colpiti da un gravissimo lutto, con un nuovo lavoratore che purtroppo ha perso la vita in occasione dei lavori nel cantiere di Capodichino. Credo che ci siano molte questioni che dovrebbero comunque attirare l'attenzione dell'Assemblea,

In verità, vorrei sottolineare l'importanza della figura dei senatori a vita, perché essi sono una componente fondamentale del sistema politico italiano.

infatti vederlo sotto vari aspetti: *in primis*, sono garanti della continuità istituzionale, perché i senatori a vita nominati per meriti speciali rappresentano una continuità storica e culturale; la loro presenza assicura che le istituzioni italiane siano radicate nella storia e nei valori della Repubblica. Proprio perché sradicati dalle dinamiche politiche, hanno un significato particolare, di cui dovremmo fare tesoro.

la nomina dei senatori a vita permette di conoscere e valorizzare il contributo dei cittadini italiani che si sono distinti i vari campi, quindi non solo è un incentivo a far sì che certe persone possano raggiungere

perché penso che abbia senso. I Presidenti della Repubblica naturalmente scelgono persone che hanno avuto il tempo di affermare questi altissimi meriti, tali da renderli appunto

dal punto di vista sistematico - indicare che il senatore o la senatrice a vita debbano essere una persona di età compatibile con i meriti necessari, per assurgere a questo altissimo incarico, a noi sembra una

Presidente, mi dispiace attirare l'antipatia del Presidente del mio Gruppo, il Gruppo Misto, ma anche... PRESIDENTE. Potrebbe alternarsi, però, non è detto: di solito, all'interno dei Gruppi,

che sia lesivo della saggezza del Capo dello Stato prevedere una soglia minima sotto la quale non nominare senatori a vita. Quindi, noi non riteniamo che l'esistenza di una soglia minima o di soglie di età possano in qualche modo determinare una maggiore saggezza ed una ponderazione che invece devono essere affidate al Capo dello Stato in quanto tale. C'è poi un elemento fondato, che illustrava prima il collega, senatore Scalfarotto, che va valutato. Evidentemente, con le aspettative di vita che aumentano, è chiaro che quando si nomina un senatore a vita che ha un'età più bassa, questi dovrò avere una valutazione ancora più ponderata, perché è evidente che questi potrà svolgere questo ruolo fino al termine dei suoi giorni. Proprio perché non riteniamo che ci debba essere una soglia sotto la quale o sopra la quale si possa essere nominati senatori a vita, noi riteniamo che già il testo costituzionale così com'è non dovrebbe essere toccato: il testo che, purtroppo, la maggioranza vuole toccare, rappresenta

intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento, volendo innanzitutto porre, di fronte all'attenzione di quest'Aula e di tutti noi, un fatto abbastanza triste e paradossale che sta accadendo durante queste ore di discussione. Siamo di fronte al silenzio dei parlamentari della maggioranza. Sì, qualche intervento c'è stato: il presidente Pera, il relatore. Ma l'obiettivo pare essere, sempre più, quello di voler accelerare i tempi, quello di voler in qualche modo comprimere la discussione e un dibattito proficuo. Colleghe e colleghi, io davvero vi vorrei invitare alla riflessione rispetto a quello che stiamo facendo. La materia che stiamo trattando è talmente delicata e importante che, non solo per il rispetto per quest'Aula, ma anche per il rispetto verso i cittadini, noi vi dovremmo dedicare il massimo dell'attenzione. Dovremmo, infatti, avere la consapevolezza che, se questa riforma dovesse essere approvata, cambierà radicalmente

figlia della Resistenza e della lotta di liberazione, è stata scritta per garantire un sistema di pesi e contrappesi, in modo da prevenire l'accentramento del potere, in modo da costruire un modello parlamentare in cui la nostra Repubblica assicura che il potere esecutivo sia bilanciato dal controllo parlamentare e dall'azione profonda del Presidente della Repubblica. Questo equilibrio è cruciale per evitare derive per fare in modo che qualsiasi decisione governativa sia davvero il frutto di un processo democratico e condiviso. Non è così con il premierato. Il premierato concentra il potere decisionale nelle mani di una sola persona, riducendo il ruolo del Parlamento,

delle sue prerogative e delle sue competenze e legato al destino di una sola persona o di un solo *leader*. Voi potreste dire: ma voi parlate così perché siete animati da uno spirito conservatore e non volete che nulla cambi. Non è così. abbiamo sempre posto l'esigenza di poter aumentare i poteri del Presidente del Consiglio, ma lo abbiamo fatto in modo diverso, per esempio attraverso la sfiducia costruttiva o indicando una strada di garanzie e di equilibrio costituzionale che non sia quella della deriva plebiscitaria e della mitologia decisionistica da parte di qualcuno. Anche qui questa mattina si è fatta una discussione relativa al fatto che

dobbiamo modificare un'architettura di fondo che garantisce l'equilibrio costituzionale. Il bipolarismo sarà poi figlio di quello che sapranno fare le forze politiche e l'alternanza non sarà la condizione di questa riforma, ma una sua conseguenza, sarà il frutto di una legge elettorale. Per tutte queste ragioni noi pensiamo che voi stiate facendo ancora una volta un errore causato dalla confusione, dall'inadeguatezza, da un certo pressappochismo: soltanto che questa volta il vostro errore ha a che fare non con il redditometro, non con l'eurobonus *(Applausi)*, non con tante altre cose di cui vi siete occupati con grandi difficoltà nel corso di questi giorni, ma ha a che fare con la carne viva dei nostri cittadini, della nostra storia e con la nostra Costituzione.

va ad abrogare una parte che noi riteniamo molto importante e che abbiamo inserito all'interno della normativa che regolamenta l'istituto dei senatori a vita, ossia quella che ne limita il numero a a cinque. Ci è sembrata questa la cosa più ragionevole per non incorrere in quel populismo becero in cui invece questa maggioranza vuole assolutamente proseguire: lo fa andando a colpire i poteri del Presidente della Repubblica di nominare cittadine e cittadini che si siano particolarmente distinti per meriti e, quindi, consentendogli di arricchire questa Assemblea con il loro contributo. Noi questo non l'abbiamo voluto fare: questa maggioranza, invece, macchiandosi del populismo più becero, vuole andare a colpire i poteri del Presidente della Repubblica. *(Applausi)*. Mi permetto però di dare un suggerimento a questa maggioranza, cercando di elevare

Se volete essere sinceramente e autenticamente populisti nel senso bello del termine, fate dimettere una Ministra che occupa quello scranno in maniera indebita. Grazie!

a tutti, anche e soprattutto ai senatori di maggioranza. Se infatti ci sarà una risposta a questa domanda, anche loro potranno dire di votare una riforma con consapevolezza, con cognizione di causa. Se la risposta invece non ci sarà, onorevoli colleghi, onorevole colleghe, voi voterete un testo,

che produrrà una sicura illegittimità costituzionale, perché il testo,

questa è la formula - un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle due Camere. Pertanto, il testo votato in Commissione prescrive al legislatore ordinario, che approverà la legge elettorale, di predisporre una legge elettorale che garantisca alle liste collegate al Presidente del Consiglio eletto una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere. Se le parole del relatore sono pronunciate con cognizione di causa, conosce qualcosa che noi probabilmente non abbiamo potuto conoscere, cioè

come sarà possibile rispettare il precetto costituzionale che voi avete proposto e votato in Commissione e che state per votare in Aula, con una legge elettorale che mette in conto l'eventualità che le liste collegate al Presidente del Consiglio eletto non raggiungano una percentuale tale da rendere possibile, con l'aggiunta del 15 per cento, la maggioranza assoluta. Se voi non siete in grado di rispondere a questa domanda o se rispondete dicendo che volete soltanto rispettare i princìpi consolidati della giurisprudenza costituzionale ed evitare quindi che ci sia un'eccessiva disproporzionalità, allora dovete riscrivere il testo della riforma costituzionale, perché esso prevede invece che al Presidente del Consiglio eletto consegua l'attribuzione alle liste collegate almeno della maggioranza assoluta. Le due cose insieme non possono stare: o la legge elettorale violerà il testo della Costituzione che voi vorreste introdurre o la legge elettorale violerà i princìpi consolidati della giurisprudenza costituzionale. *Tertium non datur,* a meno che voi non abbiate partorito una geniale idea che risolva questa aporia: ma se è così, che cosa aspettate a farcene partecipi? Che cosa aspettate a condividerla, almeno con i senatori che sono qui in Aula chiamati a difendere un testo, il cui significato non è al momento del tutto intellegibile? Pertanto, signor Presidente, rivolgo un appello, non solo al relatore e al Governo, a dirci qual è il contenuto di questa legge elettorale che dovrebbe magicamente risolvere questa contraddizione. Mi rivolgo ai senatori di maggioranza: fate valere le vostre prerogative di senatori, pretendete anche voi di conoscere ciò che state per votare nei suoi effetti. effetti. Noi stiamo discutendo di un testo del quale non riusciamo a capire fino in fondo quali effetti produrrà, nel rapporto tra Presidente del Consiglio e composizione del Parlamento.

abbastanza indiscutibile. Leggerò, in modo che i colleghi capiscano di che cosa stiamo parlando. Nel nuovo testo costituzionale che viene proposto ci sarà scritto, se dovesse essere approvato, la legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Consiglio. Ciò che diceva il presidente Balboni, cioè che questa riforma farà tendere a un bipolarismo molto netto

Questo significa che non è scritto da nessuna parte che quello che arriverà primo avrà un differenziale di seggi con la maggioranza assoluta riassumibile nel 15 Potrebbe accadere che il primo prenda il 25 per cento, il secondo il 22 per cento, il terzo il 19 per cento e via dicendo. Potrebbe tranquillamente succedere che, con più candidati Presidenti del Consiglio più o meno equivalenti, o comunque in una situazione in cui nessuno si avvicina particolarmente alla maggioranza assoluta, la distanza - che separa il candidato che arriva primo dalla maggioranza assoluta - sia superiore al 15 Dice dunque correttamente il senatore Giorgis: o è scritta male ed è sbagliata questa disposizione che parla espressamente del fatto che va garantita una maggioranza a chi diventa Presidente del Consiglio, oppure si immagina una legge elettorale in cui non viene rispettata ciò che poco fa il presidente Balboni ha detto, cioè che il premio di maggioranza non può essere superiore al 15 se così fosse, cioè se si desse vita a una legge elettorale in cui il premio di maggioranza fosse superiore al 15 per cento, si andrebbe contro la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che, come sapete, si è espressa in materia più volte negli anni passati. Una volta, ma in maniera molto significativa, ha detto che la quota riservata al premio di maggioranza non può eccedere la somma di cui stiamo dicendo. Siccome il tema che ha posto il senatore Giorgis - e che sto ponendo anch'io adesso - ci pare francamente rispondere a un elemento logico difficilmente discutibile,

le parole sono da questo punto di vista inequivocabili e nulla può portare addirittura a un bipolarismo coatto per legge, cioè a imporre per legge che i candidati debbano essere necessariamente due, basta quel premio per raggiungere la maggioranza assoluta. Penso che su questo punto il Governo e il relatore dovrebbero esprimersi e spiegare, tanto e non semplicemente a questo Parlamento ma anche a chi ci ascolta e che è fuori di qui, come si intende risolvere questa evidente anomalia contenuta nella legge. Ciò dimostra anche, come stiamo dicendo da ieri (quando mi sono lamentato del fatto che avete incredibilmente espresso un parere negativo sull'ordine del giorno del che sarebbe stato nettamente più logico discutere insieme della riforma costituzionale e della legge elettorale. In questo modo, un caso come questo, evidente e clamoroso, almeno l'avremmo potuto affrontare capendo di che cosa stavamo parlando. Invece no, ragioniamo al buio; anzi, peggio che al buio: siccome le riunioni di caminetto si fanno sempre, ma anche le riunioni riunioni di partito (vengo da quella storia, quindi non ho nulla da eccepire su questo), il fatto che qualcuno sappia più o meno come si pensa di immaginare la legge elettorale, e che però tutti gli altri non lo sappiano,

riforma del 2020, che stabilisce effettivamente quanti senatori a vita possano sedere contemporaneamente in quest'Aula. Dunque riterremmo sconveniente o comunque controverso un voto diverso da quello contrario. Vorrei aggiungere qualche osservazione. Stiamo parlando, se non altro, di una buona idea, quella rappresentata

ovvero quella di poter presentare le proprie dimissioni, oltre a quella, già vigente, di poter non accettare l'incarico nel momento in cui viene loro proposto. Questo - a nostro avviso - rappresenta un buon istituto, ma è meramente

alle votazioni di emendamenti all'articolo 1. Si parla di soppressione, di fatto, dell'istituto della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. Le note della relazione Le note della relazione illustrativa che accompagna questo testo presentano la scelta di revisione costituzionale, in particolare la soppressione di questa possibilità, come un intervento inevitabile nella prospettiva di una stabilità delle maggioranze, data l'intervenuta riduzione del numero dei parlamentari. Ora mi domando in che modo effettivamente renda più stabile la tenuta delle maggioranze l'inesistenza, in un secondo momento, di senatori a vita. Non mi sembra che ci sia un'attività parlamentare così ricca

si è complimentato più volte con la Presidenza del Consiglio. Questa condizione di fatto va a rafforzare la maggioranza in essere, totalmente in contrasto con quanto leggo nel testo delle note distribuito in Aula. Aula. Mi spiace che non sia al momento presente la ministra Alberti Casellati, che propone la soppressione di questo istituto, perché - sempre nelle note, molto interessanti e da approfondire

questo istituto, un po' controverso nella fase di discussione da parte dei nostri Padri costituenti, in fin dei conti venne introdotto tramite la proposta che venne, nell'ottobre del 1947, da Antonio Alberti. Antonio Alberti propose l'istituto; Alberti Casellati elimina ed abroga lo stesso istituto.

perché ci pare ultroneo. I senatori a vita sono senatori e immagino che si applichi loro il Regolamento del Senato, faranno tutto quello che possono fare gli altri senatori, compreso dimettersi; in quel caso le dimissioni saranno votate dall'Assemblea. Approfitto dell'occasione che mi è data per completare il ragionamento che facevo in precedenza sul bipolarismo coattivo, al quale si riferiva il senatore Balboni nel suo intervento precedente. precedente. Come accennavo in precedenza, la complessità dei fenomeni che ci troviamo ad affrontare in questo scorcio di secolo è tale da da rendere veramente difficile la sintesi tra anime politiche, sebbene compiuta in modo forzoso. Infatti, sebbene il senatore Balboni dicesse «ci dovreste fare quasi un monumento, perché vi costringiamo a stare insieme», io dicevo che in realtà anche quella coalizione di maggioranza che sembra così coesa poi, in realtà, così coesa non è. Ci sono moltissimi Non ne citavo però uno, che è particolarmente rilevante per il nostro dibattito: la legge elettorale. Oltre al superbonus, oltre alla leva obbligatoria, oltre all'Ucraina, oltre a molte altre cose, la realtà dei fatti è che noi non stiamo discutendo in questa sede della legge elettorale, sebbene la legge elettorale venga di fatto costituzionalizzata surrettiziamente nel testo di legge in esame. Nel momento in cui c'è un riferimento esplicito al meccanismo elettorale dentro il testo che stiamo votando, non ci potete non dire quale sarà la legge elettorale che si applicherà, perché state chiedendo al Parlamento di votare sostanzialmente alla cieca. Noi votiamo su un meccanismo che prevede un premio di maggioranza, ma non sappiamo qual è questo meccanismo. Come facciamo ad esprimere un'opinione, se non sappiamo di che cosa stiamo parlando? sarebbe molto utile, perché io ponevo un interrogativo: come si arriva a una sintesi dentro un mondo così complesso, come si fa a creare situazioni nelle quali ci si possa coagulare intorno a due polarità? l'uovo di Colombo, la soluzione che è davanti ai nostri occhi è che l'unica modalità - in cui davvero democraticamente si può incoraggiare il coagularsi di diverse posizioni intorno a due polarità è la legge elettorale a doppio turno col ballottaggio. È lì che l'elettore ha la possibilità di esprimere le proprie differenze, di esprimere la scelta per il candidato più vicino o per il partito più vicino alle proprie inclinazioni, alle proprie idee, alla propria visione del mondo. Poi, per ragioni di governabilità, che pure è un valore che va perseguito, all'elettore si dice «bene, tu hai ottenuto la tua rappresentatività attraverso l'espressione del voto al primo turno, adesso vieni chiamato ad esprimere una valutazione che ha più a che fare con la governabilità che con la rappresentanza, quella di scegliere, tra i due rimasti, quale sia la la persona, il candidato o la candidata che preferisci». È il meccanismo che conosciamo nei Comuni con più di 15.000 abitanti e non è un caso che sia un meccanismo prezioso, ma sotto attacco da parte di questa maggioranza, perché un pezzo della maggioranza vorrebbe estendere dalla Sicilia estendere dalla Sicilia il meccanismo al 40 per cento. E questa divisione all'interno della maggioranza c'è ancora in questo momento ed è la ragione per la quale la maggioranza, all'apparenza così coesa, e mette il Parlamento in una posizione difficile, quella di votare per un testo costituzionale a cui manca un pezzo. Per cui ci chiedete di votare sulla fiducia,

ci offre la possibilità di richiamare l'attenzione della maggioranza su un fatto che abbiamo più volte segnalato in Commissione, totalmente inascoltati. La maggioranza ha cominciato a discutere della questione della legge elettorale da accompagnare alla riforma costituzionale e su come tradurla in norme partendo da un presupposto che non sta in piedi, come più volte abbiamo cercato di far comprendere alla maggioranza stessa. Qual è il presupposto dal quale la maggioranza è partita?

Ma la trasposizione a livello nazionale del modello di governo dei Comuni e anche del modello di legge elettorale dei Comuni non è possibile - come abbiamo più volte spiegato - per la semplice ragione che a livello statale, le Camere, le assemblee legislative, non sono una, ma due, e il Parlamento, a differenza dei consigli comunali, è un potere dello Stato; in Costituzione cioè precisato come dev'essere composto, quali funzioni ha e secondo quali regole deve funzionare. Niente di tutto questo esiste per i consigli comunali. Il modello che nei Comuni sopra i 15.000 abitanti - come richiamava poc'anzi il senatore Scalfarotto - consente di fare il trascinamento del consiglio comunale rispetto alle elezioni del sindaco, ma con la soglia al 50 per cento, senza

elettorale comunale ha comunque dovuto prevedere. Il primo caso è quello nel quale la maggioranza del sindaco sconfitto abbia conseguito più del 50 per cento dei voti al primo turno; il secondo caso, più raro ancora, è quello in cui ci sia qualcuno eletto al primo turno, ma con la sua compagine di liste sotto il 40 per cento. Sono due casi che si sono verificati pochissime volte. In generale, nei Comuni il meccanismo del trascinamento funziona: l'elezione della persona, cioè, si porta dietro la maggioranza. che evidentemente hanno in testa coloro che hanno provato a scrivere queste norme non funziona assolutamente a livello nazionale, però, perché sono troppe le differenze e perché c'è il bicameralismo paritario. Siete quindi caduti vittima delle vostre macchinazioni e siete caduti vittima del fatto che non ci volete ascoltare, qualsiasi cosa diciamo: neanche quando diamo un consiglio con finalità del tutto trasparenti. Siamo contrari all'elezione diretta: che convenienza avremmo dal suggerirvi il modo per renderla funzionante? Pensateci bene: non avremmo alcuna convenienza dal suggerirvelo, eppure il senso di responsabilità istituzionale ci porta ad avvertirvi, anche se non siamo favorevoli all'elezione diretta, diretta, che così come la volete fare non sta in piedi. E infatti siete entrati nel caos e i vostri interventi in Aula nelle ultime quarantott'ore sono la celebrazione e l'espressione massima del caos. Un po' non ce lo volete dire, che legge elettorale farete in accompagnamento alla riforma costituzionale; ma soprattutto non ne avete la più pallida idea, perché - come vi ha detto il senatore Giorgis o violate la riforma che avete appena scritto con il verbo «garantire» o violate le sentenze della Corte costituzionale o dovete far finta che il bicameralismo paritario non ci sia. Ma il bicameralismo paritario è vivo e lotta insieme a voi e anche a noi.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, l'emendamento che proverò a difendere e che porta la mia prima firma torna a incidere sulla rilevante questione dei senatori a vita e sulla espropriata prerogativa del Presidente della Repubblica di nominarli. Nel distico che spiega il senso etimologico, che dispiega la prerogativa del Presidente, il senatore a vita è colui che ha illustrato, dunque illuminato, portato lustro alla Patria. Come preferibile, quanto profonda la parola Patria è rispetto alla più cupa Nazione; parola della quale la destra, che si balocca con l'identità, fa un uso smodato fino alla ridondanza, alla insignificanza, alla irrilevanza.

Nazione. Senatore a vita è chi ha dato lustro alla Patria per i suoi altissimi meriti: notare il superlativo. Ecco un'altra parola di cui la destra al potere fa un uso peculiare, tanto da averci addirittura intitolato un Ministero, nella sua *vis* nella sua *vis* palingenetica, di rifondazione di una neolingua, ad inaugurare, da antica tentazione, una nuova era. Signor Presidente, dicevo degli altissimi meriti dei senatori a vita in campo sociale, scientifico, artistico, letterario; insomma, meriti che il Governo vanta per il dicastero guidato dal Ministro dei dinosauri - il Ministro che rappresenta gli italiani e giura sulla Costituzione, ma porta sul bavero la spilletta di Alberto da Giussano, come fosse un militante e non un Ministro - che valgono per il Ministro dei dinosauri, non valgono per i senatori

vendetta contro i senatori a vita, che - come detto - costituisce un attacco non solo contro loro, ma anche contro il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Il punto è che non si capisce davvero cosa abbiate da temere dalla presenza in Aula di queste cinque persone. Ne temete il confronto, come se il raffronto con i loro successi, con le loro affermazioni professionali, prima evocate dal senatore Gasparri, con la loro chiara fama, possa diminuire il vostro lavoro, la vostra reputazione, il vostro profilo? Non sopportate, dunque, la loro eccellenza, che fa ombra? Oppure ciò che non va giù è la loro indipendenza ed autonomia di giudizio? La loro autonomia, che suona come un monito nei confronti di una politica, che *superiorem non recognoscens*, che preferisce il capo alla libertà di giudizio, che non sopporta lo scarto del pensiero, che predilige l'obbedienza, pronta, cieca, assoluta? peggio ancora, signor Presidente, è la loro autorità morale a non essere digerita? A suonare come un giudizio inappellabile, uno specchio deformante rispetto alla Camera anecoica di plausi e corriva compiacenza, che spesso i governanti cercano, bramano, premiano? Non mi è, caro Presidente, quale sia la colpa, qual è il dolo imperdonabile dei senatori a vita, di quelli di oggi e di quelli di ieri. È come se fossero una macchia nella retina di una destra che non li tollera, come non tollera il corpo estraneo, l'intruso, l'inassimilabile, l'eterodosso, l'anomalia, non diceva, il presidente Balboni. Dietro al riflesso che porta alla cancellazione dei senatori a vita, alla loro epurazione, c'è qualcosa di profondo e di oscuro che davvero inquieta il Parlamento e i cittadini che il Parlamento rappresenta. Su questo punto ci torneremo. In fondo quello che vediamo agire qui lo ritroviamo in tanti altri ambiti, in quello europeo, in una visione dell'altro, del prossimo, dell'anomalia, fatta di sospetto e allarme, di chiusura, di scarsa attitudine al confronto, alla mescola, all'accettazione della diversità come ricchezza, come patrimonio, il terzo escluso. Pensate anche da questo, forse soprattutto da questo, si vede chi siamo, chi possiamo essere, chi siamo condannati ad essere. *(Applausi)*.

Prego, nell'intervento che prima sono stato costretto a interrompere perché era scaduto il tempo, mi ero concentrato sull'indicazione dei motivi per cui non è giusto che vi presentiate - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - come difensori della

che abbia molto potere, ma contro di sé la maggioranza degli italiani, è uno dei modi con cui calpestate la sovranità popolare. La calpestate poi con la coltre di buio sotto cui avete sepolto i vostri intendimenti per quanto riguarda il modo di eleggere i parlamentari. Se non c'è chiarezza sul modo di eleggere i parlamentari, che sono coloro che compongono le due Camere, cioè l'espressione massima della sovranità del popolo, quale omaggio alla sovranità popolare c'è? C'è un agguato alla sovranità popolare, non un omaggio. L'altro motivo è quello del Parlamento eletto a strascico. Riflettiamo bene su ciò che significa in termini di difesa della sovranità popolare. Il Parlamento è il luogo delle istituzioni che, come corpo collegiale, rappresenta o meglio dovrebbe rappresentare tutte le opinioni che ci sono nel Paese in una misura rilevante. Non c'è quindi un posto dove la sovranità popolare è maggiormente rappresentata e trova maggiormente spazio e voce. e voce. Dal modo in cui si tratta il Parlamento si capisce, pertanto, qual è l'opinione che si ha della sovranità popolare; se davvero si dà centralità al popolo o se invece al popolo si rende un omaggio formale, cercando di fregarlo sottobanco. È abbastanza evidente che voi questo popolo, che formalmente omaggiate, in realtà sottobanco cercate di fregarlo. Il Parlamento oggetto di un'elezione ancillare, ausiliaria, subordinata, che è il sottoprodotto di un'elezione di una persona, non c'è in alcun posto del mondo, nemmeno nel più sbilanciato e squilibrato sistema presidenziale del pianeta. Dovunque il potere legislativo è o prevalente rispetto a quello esecutivo o è, in parallelo con l'esecutivo, autonomo e indipendente. In nessun Paese del mondo il Parlamento è a ruota di una persona o del Governo, sottoposto e asservito formalmente al potere esecutivo. Vi state mettendo su una strada che non è brutta soltanto perché rappresenta un *unicum* mondiale, ma perché è anche il rovesciamento completo dei princìpi che guidarono i nostri Padri costituenti nell'organizzare il rapporto tra i poteri dello Stato. Ripeto: queste cose fanno capire che gli scappellamenti verso la sovranità popolare sono un grandissimo atto di ipocrisia con cui cercate di gettare fumo negli occhi dei cittadini. In realtà alla sovranità popolare assestate dei colpi gravi, che noi cercheremo in qualsiasi modo di parare nell'interesse del Parlamento e dei cittadini italiani.

di quello che abbiamo provato a dire - ma la ministra Casellati naturalmente lo sa bene e lo sa bene anche il presidente Balboni - molte volte in questi mesi di discussione in Commissione. A me davvero spiace che sia stato preso come un atteggiamento preconcetto

Mi dispiace doverlo dire, ma il solo fatto che da parte dei banchi del Governo o della maggioranza non si intervenga - e non si dica che non è vero, che ci stiamo sbagliando perché le cose stanno così e non stanno come diciamo noi - è proprio indicativo del fatto che evidentemente, invece, quello che le forze dell'opposizione stanno sostenendo ha un fondamento: c'è una palese contraddizione tra l'articolo così come l'avete scritto, le sentenze della Corte costituzionale e la dichiarazione che ha fatto poco fa il presidente Balboni quando parlava espressamente di un premio di maggioranza non superiore al 15 per cento. Queste cose non si tengono, ve lo stiamo dicendo più volte oggi e ve lo abbiamo detto in Commissione tante volte. Tuttavia, non ci rispondete e le mancate risposte ci fanno capire chiaramente che, almeno su questo punto, siamo dinanzi a dinanzi a un cortocircuito e che probabilmente anche tra le forze di maggioranza, allo stato attuale, non c'è un accordo o comunque non c'è una soluzione rispetto a questo problema dato. Tuttavia, per fare una considerazione politica e non ripetere quanto ho detto nello scorso intervento, questa vicenda da sola dimostra davvero molto chiaramente come la propaganda si ferma davanti alla realtà. Per esempio, parlare - come purtroppo è stato fatto in tutti questi mesi - del sindaco d'Italia, come se si potesse esportare il modello che si usa nei consigli comunali allo Stato, facendo finta che i Comuni, le Regioni e lo Stato non siano cose differenti, probabilmente - come ben si vede - è stato un errore. Le semplificazioni non servono, non portano da nessuna parte: i Comuni sono gli enti dove si discute, giustamente, seriamente e legittimamente dei piani regolatori, quindi di cose serissime, naturalmente, per carità, quindi probabilmente desta meno scalpore un effetto trascinamento. Io vivo in una città nella quale una decina d'anni fa, la prima volta che Luigi de Magistris divenne sindaco di Napoli, aveva preso al primo turno - mi sembra,

che avevano preso le liste al primo turno si trasformò nel 60 per cento dei seggi. Quindi liste che avevano ottenuto il 12 per cento dei voti dei cittadini napoletani avevano poi preso

si portò con sé un enorme effetto trascinamento che moltiplicò i seggi delle liste per sei volte. Pensate voi che clamoroso trascinamento!

comunali non si elegge il Presidente della Repubblica, non si eleggono i giudici della Corte costituzionale, non ci sono i processi di revisione costituzionale. L'amministrazione di

Comuni, Province, Regioni, Stato nella sciagurata modifica del Titolo V della Costituzione; però, come ben si vede, immaginare di trattare la forma di governo dello Stato come se fosse un Comune è un enorme errore politico. diciamo che, con un ruolo non particolarmente attivo della maggioranza in questo dibattito, un po' ce la cantiamo e ce la suoniamo. Voglio quindi ribattere alle cose che ha detto il mio stimatissimo collega De Cristofaro, con il quale su questo ho un'opinione abbastanza divergente e che era poi la ragione della nostra apertura di credito nei confronti della ministra Casellati e del suo sforzo. io rivendico l'espressione "sindaco d'Italia", perché sarà pure una semplificazione, ma è fuori discussione che il modello di governo dei sindaci, il modello di governo dei Comuni con più di 15.000 abitanti, è il modello istituzionale di amministrazione, in questo caso - che funziona meglio e in cui di più si riconoscono i nostri concittadini. Il sindaco è un personaggio riconoscibile: è il capo di una comunità, è eletto con un sistema a doppio turno, e quindi è sempre il sindaco della maggioranza assoluta dei cittadini. L'esperienza di questi ormai molti anni, nei quali abbiamo utilizzato questo sistema, ci dice che i sindaci italiani sono tra le figure istituzionali più riconoscibili e più stimate, e che la distanza che si misura tra l'elettorato e il proprio Comune di appartenenza è forse la minore se guardiamo al rapporto tra i cittadini e le varie istituzioni della Repubblica. Pertanto, allargare quel sistema, nel senso di individuare un capo dell'Esecutivo che sia immediatamente riconoscibile, che sia scelto con voto dei cittadini, che abbia poi ovviamente anche la possibilità di governare per l'intero periodo per il quale è stato chiamato a svolgere quell'incarico, noi pensiamo sia qualcosa che

e si esaurisce con un Governo di unità nazionale presieduto - secondo me fortunatamente per il nostro Paese - dal presidente Draghi: un esito completamente diverso da quello che il corpo elettorale ci aveva dato nel 2018. Per questo noi diciamo che è necessario arrivare a una riforma costituzionale. Il distacco tra l'elettorato e le istituzioni è dovuto anche al fatto che, una volta che si è votato, l'effetto di quel voto è completamente staccato dalla sua causa: il voto va in una direzione e la politica e le istituzioni vanno in una direzione completamente imprevedibile. Questo non può funzionare. Parlare però di sindaco d'Italia non significa pedissequamente applicare un modello a un contesto che, come dicevano i colleghi Parrini e De Cristofaro, è oggettivamente diversa da un Comune. È chiaro che il Parlamento ha tutta una serie di caratteristiche che lo differenziano, ma questo non ci avrebbe dovuto impedire di provare ad adattare quel modello alle specificità del Parlamento. Visto che noi qui, da legislatori anche costituzionali, abbiamo una pagina bianca davanti, nulla impediva alle forze politiche, condiviso l'obiettivo, di scrivere insieme una riforma che tenesse conto delle specificità del Parlamento nazionale, ma che conservasse

è perché neanche la maggioranza è d'accordo al proprio interno su tale questione. È la ragione per la quale noi discutiamo di un sistema elettorale evocato dalla Costituzione, ma del quale nessuno sa nulla.

nel dibattito tra il senatore De Cristofaro e il senatore Scalfarotto al riguardo del sindaco d'Italia. Ricordo al senatore Scalfarotto - per il suo tramite, Presidente - che il consiglio comunale ha però un'ulteriore possibilità, ossia un contrappeso: far dimettere il 50 per cento più uno dei consiglieri comunali e far comunque cadere il sindaco. Quindi non è il viceversa in cui abbiamo un sindaco che si dimette, si va tutti a casa e basta; abbiamo anche il contropotere, nel momento in cui ci fosse una una deriva da parte del sindaco, che si distacchi dalla propria maggioranza. Detto questo, mi sia consentito anche rispondere al presidente Balboni, che prima ha citato un articolo di «PublicPolicy» relativamente a una dichiarazione del senatore Crimi riguardo all'abolizione dei senatori a vita. Ricordo che il senatore Crimi propose sulla nostra piattaforma alla tutti i nostri iscritti, la possibilità di proporre un disegno di legge che appunto portasse all'abrogazione dei senatori a vita. Siccome non tutti i parlamentari e non tutti gli iscritti erano d'accordo su quella proposta, ci fu una votazione. Noi ci teniamo alla nostra democrazia interna e, laddove non si sia tutti d'accordo, facciamo votare gli iscritti. È banale: facciamo votare gli iscritti. *(Applausi)*. Io mi chiedo come facciate voi, invece, al momento delle decisioni, perché a me risulta che decida tutto la famiglia Meloni. Avete un Ministro, avete il Primo Ministro, avete il capo segreteria del partito: è tutto in mano alla famiglia. *(Applausi)*. A me non sembra che sia poi così democratico il vostro partito. Detto questo, rispondo anche al senatore De Carlo, che prima, con una battuta fuori microfono, ha detto «licenziate Crimi». Vede, senatore De Carlo - sempre per il suo tramite, Presidente - noi chi la pensa diversamente non lo buttiamo fuori. Noi buttiamo fuori chi si occupa della cosa pubblica in modo disonesto. Ed è quello che voi non fate, nonostante abbiate un codice etico e comportamentale che dovrebbe vietare di avere Ministri gravemente rei di comportamenti rei di comportamenti apparentemente disonesti, anche se non ancora condannati. Il vostro codice etico prevede comunque che siano sospesi: ma voi, allo stato attuale, non lo avete fatto. Quindi dare lezioni di democrazia al MoVimento 5 Stelle mi sembra fuori da ogni logica da parte di Fratelli d'Italia. Sempre il Sempre il presidente Balboni prima diceva che si tende o si auspica che questo porti a un bipolarismo. Mi auguro che non sia in senso clinico, questa frase: ciò perché a quel punto la capirei, se fosse in senso psichiatrico. Voi state dicendo agli elettori, che già si astengono, che sarebbe giusto e corretto che, ad esempio, un elettore della Lega della vecchia scuola (quella secessionista, per intenderci) debba andare a votare quello che sarà il Presidente del Consiglio della forza politica nazionalista, che ovviamente è per tutta un'altra politica. Polarizzare sui temi, come diceva prima il senatore Scalfarotto, non fa altro che allontanare le persone dal voto, perché io non andrò mai a votare una coalizione che ha al suo interno delle forze politiche che la pensano diametralmente all'opposto di come la penso io, a meno che non mettiate il ballottaggio. A quel punto sì; sempre in disaccordo con il con il senatore Scalfarotto, aggiungo che io, da elettore che non ha votato al primo turno i due che vanno al ballottaggio, non voterò quello più vicino a me, perché l'avevo già votato al primo turno, ma andrò a votare quello meno lontano dalle mie idee, penalizzando quello che, secondo i miei valori, meno mi rappresenta. È per questo che avete paura del ballottaggio, perché tutte le volte che c'è un ballottaggio il cittadino libero vota anche il meno peggio.

non ha alcun senso.

Signor Presidente, per rispetto dei Gruppi più piccoli, i cui membri non hanno la possibilità di alternarsi come gli altri, una piccola pausa sarebbe veramente

credo che realisticamente poi sarebbe difficile ricomporre l'Assemblea; non è meglio andare avanti fino alle ore 14,15 e poi anticipare la chiusura dei lavori? Sospendere e riprendere mi pare complicato per tutti.

più difficile. Questo emendamento vuole inserire un criterio di proporzionalità nell'articolo 59, ma mi rendo conto che parlare nel merito degli emendamenti è tempo perso. Mi rendo conto che questa maggioranza non ha più neppure voglia di ascoltare quello che sta dicendo l'opposizione. *(Brusio).* Colleghi, scusate, non riesco a mantenere la concentrazione. PRESIDENTE. Sì, senatore Cataldi, sto facendo fatica anch'io. Per favore, colleghi,

è l'equilibrio costituzionale, lo Stato di diritto e la divisione dei poteri. Questo è il problema dell'Italia e questa è la grande riforma, la madre di tutte le riforme. Questa stortura democratica la volete giustificare col pretesto della stabilità,

l'Italia avrà un Governo più stabile, perché la stabilità viene rimessa agli umori di una sola persona, che può decidere da un giorno all'altro di ritornare al voto senza che nessuno possa dire nulla, nemmeno il Presidente della Repubblica? Ma quale imprenditore sarà così folle da investire in un Paese così? Quale imprenditore farà *business* in Italia, sapendo che una sola persona può decidere la stabilità del Paese? però avete inserito anche un altro meccanismo. Supponiamo che questo *super premier* non si dimetta e non ci faccia tornare al voto, bontà sua.

inadeguato al compito, se c'è una situazione di crisi, se si dimostra incapace, se dimostra essere colluso con la criminalità organizzata, il Parlamento non lo sfiducerà, non perché farà una scelta onesta, ma perché voi riponete la stabilità sulla illusione che i prossimi parlamentari preferiranno scelte conservative. Quindi, voi pensate che la stabilità dipenda dalla disonestà dei parlamentari che, invece di mandare a casa un *premier* disonesto, sceglieranno di mantenere il posto e continueranno ad appoggiarlo. Vi sembra questo il modo di garantire la stabilità? Se i parlamentari, come sono convinto, saranno onesti, voi state invece creando una doppia instabilità, perché, non soltanto se ne andrà il *premier*, ma cadrà anche il Parlamento. non create nessuna stabilità. Sapete quale stabilità state creando? Voi state stabilizzando l'usurpazione del potere legislativo, perché non avete voluto accogliere un emendamento della senatrice Maiorino sull'articolo 77. Quindi, voi darete

della Costituzione, quindi il tema dei senatori a vita. Io capisco che, anche in quest'Aula, dedicare così tante ore a parlare del ruolo, della funzione e dell'importanza dei senatori a vita può apparire, per alcuni colleghi, quasi un tentativo ostruzionistico.

Qui l'opposizione non sta mettendo in atto delle misure che stiano limitando in qualche modo la maggioranza. La scelta dell'opposizione, con la presentazione di tanti emendamenti sullo stesso tema, è nata dal fatto di voler discutere anche in Aula. Io non sono membro della 1ª Commissione, ma ho partecipato ad alcune sue sedute. Sostanzialmente, anche il presidente Balboni non potrà smentire che gli interventi dell'opposizione sono stati molto numerosi rispetto a quelli della maggioranza, che ha

in riforme così importanti, la maggioranza è sempre stata protagonista delle riforme, facendo in modo che il dibattito in Commissione e in Aula, anche grazie agli emendamenti, fosse ricco. Abbiamo capito, però, che non è questo questo il tempo. La maggioranza qui ha deciso di far coincidere esattamente la propria volontà con quella del Governo e quindi ha rifiutato di svolgere questo ruolo. Voglio, però, ritornare su quello che viene definito ostruzionismo, perché io ritengo che la necessità di evidenziare così tanto emendamenti rispetto ad una stessa materia nasca dal fatto di voler provare a stimolare una qualche discussione con tutta una serie di varianti. È come se l'opposizione avesse presentato, attraverso questi emendamenti, una serie di possibilità alla maggioranza, dicendo: se volete toccare esattamente quell'articolo, ci sono tante sfumature con cui poterlo affrontare, mantenendo però - dice l'opposizione - chiaro un principio in tutti gli emendamenti: che i senatori a vita in qualche modo devono rimanere. Ma perché devono rimanere? In quest'Aula ci sono stati colleghi dell'opposizione che hanno svolto interventi meravigliosi e che sarà anche un piacere rileggere negli anni a venire. Io non svolgerò un intervento di questo livello, ma ci tengo a lasciare traccia del perché sia importante mantenere l'articolo con quelle caratteristiche.

con due Camere che non erano esattamente uguali; il Senato cambiava per bacino elettorale, in quanto veniva eletto da un bacino diverso rispetto a quello della Camera per quanto riguarda l'età e si può accedere con un'età diversa. Si era cercato così di non renderle esattamente coincidenti proprio per la necessità che, in un sistema come quello parlamentare italiano, ci fosse un elemento aggiuntivo.

La prego di concludere, senatrice. lasciare traccia di una diversità, proveniente però dal mondo esterno. Se vuole, Presidente, è quello che noi siamo chiamati a fare e dovremmo fare

La mia paura, allora, visto che in questo ultimo anno e mezzo la stiamo proprio vivendo così, è che anche questi mondi esterni non vengano più considerati importanti: che vengano chiamati in audizione e, poi, non ascoltati. La malattia di cui questa maggioranza vive è infatti quella di pensare di essere autosufficiente, di non aver bisogno di nessuno. La politica, però, quando pensa...

ha parlato di quasi ostruzionismo. Ha ragione, in realtà questo è un quasi ostruzionismo, che poi francamente impallidisce rispetto all'ostruzionismo così com'era una volta. L'ho detto anche in Commissione; basta

Il segretario del Movimento sociale Giorgio Almirante parlò per nove ore consecutive contro lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Sono cose che sappiamo e quindi non c'è bisogno di sottolinearle. In realtà ha ragione la senatrice Malpezzi a definirlo quasi ostruzionismo. Ciò ha a che fare con la discussione che facciamo in queste ore.

che l'ostruzionismo parlamentare, molto utilizzato da alcuni partiti politici di opposizione nel corso della cosiddetta Prima Repubblica, sbilanciasse eccessivamente i rapporti di forza a favore del Parlamento e quindi bilanciasse l'iniziativa legislativa del Governo con l'iniziativa del Parlamento. Non è un caso che l'ostruzionismo è stato ridotto nel corso degli anni. Non è mica una cosa figlia del destino: ha avuto a che fare con un preciso indirizzo politico-culturale che si è sviluppato da molti anni a questa parte, teso a puntare esattamente su questo punto, cioè sull'idea che bisogna dare più poteri al Governo e meno al Parlamento, perché bisogna favorire la stabilità. Insomma, sono esattamente le stesse cose che sentiamo oggi. Faccio queste osservazioni in riferimento alle parole che stiamo ascoltando, almeno che io sto ascoltando da molti mesi anche in Commissione, a questa sorta di ossessione per la stabilità. Non voglio sminuire la stabilità, perché capisco anch'io che è meglio avere qualche Governo in meno e che non è proprio il massimo della vita cambiare un Governo all'anno; ma questa ossessione della stabilità è stata esattamente il centro propulsore attorno al quale ha ruotato un pezzo ampio di dibattito politico e istituzionale da molti decenni. Questo è l'ultimo frutto di una lunga stagione politica. Ma è esattamente questa la ragione per cui vi chiedo perché non si prova a fare un bilancio, non di questi sei mesi di riforma Alberti Casellati, ma di questi quarant'anni. Si provi a fare un bilancio dell'intera storia della Seconda Repubblica, cominciata quando con Tangentopoli cadeva nelle macerie la storia della Prima Repubblica, quella dei partiti, quella dei corpi intermedi: cominciava una stagione politica diversa, segnata da leggi maggioritarie, dai partiti personali, dai nomi dei *leader* nei simboli di partito, quello che è successo negli ultimi trent'anni. La cosa che a me sarebbe piaciuta, in questo caso più più che come senatore della Repubblica anche semplicemente come cittadino interessato alla cosa pubblica e alle dinamiche politiche, sarebbe stato esattamente capire se, dinanzi a questi processi, l'indirizzo politico scelto in questi decenni ha accentuato alcuni elementi di crisi oppure li ha risolti. Siccome io faccio parte di quelli che pensano che questi elementi di crisi sono stati profondamente accentuati da questo indirizzo politico-culturale, avrei trovato molto intelligente fare un bilancio di questi decenni e capire anche se era possibile invertire la tendenza. Invece, purtroppo, si va esattamente nella stessa direzione, con l'orchestra che suona senza vedere che davanti c'è l'*iceberg* sul quale, purtroppo, rischia di sfracellarsi la Repubblica italiana.

senatori a vita. Il ricordo che mi si è sbloccato questa notte è che l'11 dicembre 2013 la Giunta per le elezioni del Senato ha convalidato l'incarico di senatori a vita nominati dal Presidente Napolitano, ossia Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia.

all'istituto». Ecco perché al ricordo sbloccato si è aggiunto il ricordo sonoro di una canzone bellissima che dice: «Come si cambia, per non morire». devo anche dire che le ragioni che all'epoca il Movimento 5 Stelle, che diceva ancora quello che pensava e faceva quello che diceva, erano che i senatori a vita potevano in qualche modo influire sulla vita del Parlamento, soprattutto del Senato, democraticamente eletto. È quello che noi diciamo oggi, ancor di più mettendo in evidenza quello che è stato giustamente detto prima, ossia che non abbiamo notizie di scienziati, artisti, cultori di un'area politica nominati senatori a vita. Quindi pensiamo che, con questi pochi numeri del Senato, i senatori a vita potrebbero in teoria dirimere o indirizzare in un modo o nell'altro i voti di fiducia. Noi siamo rimasti della stessa idea da sempre; qualcun altro questa idea

mi dispiace per il senatore Berrino per la brutta notte che ha avuto *(Applausi)*. Penso che ci siano modi più interessanti per passare le proprie notti, anche dormendo eventualmente, senza ricorrere ad altri tipi di cene. Detto da chi doveva fare blocco navale e si piega all'Europa; da chi diceva che la pacchia è finita in Europa e si piega al Patto di stabilità; da chi diceva "mai il redditometro" *(Applausi)*e poi ha un Vice Ministro che inserisce il redditometro: ecco, «Come si cambia, per non morire» probabilmente è il prossimo slogan per Fratelli d'Italia. La questione è che questo tipo di posizione del MoVimento si inserisce - cerco di essere un po' più serio - in un quadro di modifica costituzionale che va a toccare e indebolire le prerogative del Presidente della Repubblica. È questo il motivo per cui, pur avendo avuto da sempre le perplessità e le posizioni che sono state ricordate sulla questione dei senatori a vita, riteniamo che in questo contesto andare a toccare anche quelle prerogative del Presidente della Repubblica sia profondamente sbagliato. *(Applausi)*.

colgo l'occasione di questo emendamento per tornare a un tema che già ha attraversato una parte delle dichiarazioni di voto sugli emendamenti, cioè quello che

con queste caratteristiche nel Senato della Repubblica, sarebbe un elemento di fastidio. Le spiegazioni, quelle poche che finora ci sono state date, mi paiono tutte sottrarsi alla domanda fondamentale. Perché non ci può essere un luogo in cui si riconoscono quelle caratteristiche e in quello stesso luogo noi, che siamo i soggetti

gli eletti, le figure che danno maggiore lustro al Paese e le figure che rappresentano tutte le caratteristiche della società civile e le tensioni che ci sono nel Paese? Io penso che siamo presi da un'idea

oggi il Presidente della Repubblica è quella figura che tiene insieme la relazione tra il Paese, i cittadini e le istituzioni. Nel momento in cui volete indebolire quella figura, cioè costruire una divaricazione tra l'insieme della società e le Istituzioni, è anche ragionevole che non ci siano altri soggetti che possano rappresentare quella possibilità. Ciò che però continua a non convincermi e a non essere comprensibile è perché volete fare questa operazione. Qual è la ragione che spinge ad immaginare che, in un Paese che ha sicuramente un problema di debolezza istituzionale dato dalla lontananza dei cittadini rispetto alle Istituzioni, dalla sfiducia, dal senso di non partecipazione, la risposta sia che le Istituzioni diventano ancor di più delle torri d'avorio irraggiungibili da chiunque? Credo che sia l'operazione esattamente opposta a quella di cui ha bisogno non solo la democrazia, ma anche proprio la credibilità della nostra azione politica e delle risposte che si danno. E lo dico perché tutte le volte

delle forme di rappresentanza rispetto ai corpi intermedi o alle forme di partecipazione, c'è stata una relazione netta e immediata con la partecipazione dei cittadini. Lo dico anche pensando a cose fatte da questa parte dell'emiciclo, non necessariamente a quelle che sono state fatte dall'altra parte. Adesso non raccontatemi la solita storia, perché al Governo ci siete stati anche voi ininterrottamente in tutti questi anni; quindi tutti hanno delle responsabilità.

che hanno determinato distanza tra la partecipazione delle persone e la riconoscibilità delle persone in azione, hanno determinato immediatamente un abbandono e un aumento dell'astensione alle elezioni. Proviamo a riconnettere queste due cose e a domandarci se, allora, la *ratio* che dice "noi ci mettiamo nella torre d'avorio, perché siamo in grado di decidere e di fare tutto, anche con maggioranze molto discutibili" non sia invece un ulteriore argomento usato per l'indebolimento della democrazia e della partecipazione. Oppure continuiamo a far finta che, se ce la raccontiamo tra di noi, noi, la racconta anche tutto il mondo. Purtroppo, siccome il mondo ci guarda (il mondo inteso come il nostro Paese e la nostra Nazione), ciò che rischiate di determinare è esattamente che continui a esserci una fuga dalla partecipazione. Una democrazia debole non è debole solo per l'opposizione; una democrazia debole è debole per

i cittadini si rendono conto che, mentre il Paese deve affrontare problemi gravissimi, ci sono un Parlamento e una politica che si occupano di tutt'altro e di emergenze che sono tali solo per la forza politica al Governo. Mentre stiamo qui in

che sono soprattutto giovani e quelle donne che dite di voler aiutare. Ci sono oltre 4 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi, perché non possono permettersi di accedere alla sanità privata. Ci sono 120.000 giovani che lasciano l'Italia ogni anno per non fare più ritorno, perché qui non hanno possibilità di futuro. E allora, mentre fuori c'è un Paese che aspetta queste risposte, noi qui parliamo in modo assolutamente autoreferenziale di questi pastrocchi che vi piacciono così tanto, ma che non faranno altro che rendere più complicata la vita dei cittadini.

di democrazia partecipata che continuiamo a difendere. Signor Presidente, tengo anche a raccontare un altro progetto che mi onoro di portare avanti ormai da più di un anno, che riguarda un intergruppo che si occupa proprio di parlare di diritti e che vede ogni mese riuniti qui in Senato oltre cento cittadini che si mettono a discutere assieme delle soluzioni ai problemi concreti del Paese e costruiscono proposte che sono diventate anche disegni di legge. Occupiamoci di questo e non andiamo invece a eliminare anche quell'unico spiraglio di partecipazione democratica e della società civile alla vita parlamentare che oggi è rappresentato quasi esclusivamente, oltre che da alcune forze politiche che candidano anche comuni cittadini, dalla possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita. Questi senatori a vita, come ieri abbiamo detto chiaramente, vengono nominati in base agli altissimi meriti che hanno dimostrato di avere e che sicuramente rappresentano un valore aggiunto. Vi voglio ricordare quanto soprattutto durante la pandemia, quando per la prima volta la politica ha cominciato a fare scelte leggendo anche i dati scientifici, avere in quest'Aula scienziati e persone che potevano aiutare i politici a prendere decisioni. Rivendico

privati). Ciò vuol dire che gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono i più bassi d'Europa. Nonostante questo, signor Presidente, nonostante gli investimenti siano praticamente pari a zero, i nostri scienziati e i nostri ricercatori sono ai primi posti in tutte le classifiche scientifiche perché, nonostante quei pochissimi finanziamenti, riescono a pubblicare ricerche d'eccellenza. Non ci possiamo permettere però di continuare a regalare i nostri investimenti agli altri Paesi, perché, se spendiamo 400.000 euro per formare un dottore di ricerca e poi sono pochissimi quelli che lavorano in Italia, perché gli altri vanno a lavorare all'estero, dove generano ricchezza e attraggono finanziamenti, questi sì che sono investimenti a perdere. Occupiamoci quindi di quelle che sono veramente le emergenze del Paese.

che si cambi opinione che ogni tanto cambiare opinione non fa neanche male; è capitato anche a me (poche volte, per la verità, perché sono abbastanza duro di testa):

perché è sotto gli occhi di tutti, è pensare che la semplificazione e il fatto di dare il potere in mano a una sola persona di per sé risolva il problema.

in larga minoranza, ma questa è la mia opinione e ci tengo a sottolinearla, visto e considerato che sono in larga minoranza anche nella mia formazione politica.

io sono contento che al senatore Berrino si sia sbloccato un ricordo. Egli deve, però, avere un meccanismo per cui, quando si sbloccano i ricordi, si disattiva l'attenzione. Credo, infatti, gli sia sfuggito, che da ieri, alle ore dell'emendamento 1.1002, che contiene la posizione del MoVimento, e che conferma quanto il senatore Berrino ha detto sia essere

presentato un emendamento con cui, per evitare che ci sia troppa interferenza con la maggioranza del Parlamento, si toglie il voto ai senatori a vita sulla questione di fiducia. È una cosa che denunciavamo nel 2013 e denunciamo anche ora. Quindi mi fa piacere che si sblocchino i ricordi; spero che si sbloccherà anche l'attenzione e che il senatore Berrino voterà a favore del nostro emendamento, che è esattamente quello che chiedeva lui.

il personale ATA costituisce una risorsa fondamentale e indispensabile per la molteplicità di compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica. Il medesimo personale si è dimostrato essenziale per supportare le istituzioni anche nell'attuazione dei progetti del PNRR e dell'Agenda del Mezzogiorno.

le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA sono aggiornate con cadenza triennale e sono utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee. Da una prima bozza di decreto si prevedeva l'apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande dal 20 maggio al 20 giugno, mentre successivamente si pensava che che il termine temporale fosse dal 28 maggio al 28 giugno; però ad ora non è ancora stato pubblicato un testo definitivo del decreto. Le chiedo quindi, signor Ministro, quando verrà decreto, in modo tale da dare delle risposte concrete al personale ATA, e quali azioni ha direttamente posto in essere per valorizzare queste figure. Signor Presidente, gentili senatori, condivido pienamente le parole della senatrice relativamente al carattere fondamentale del personale ATA per la nostra scuola davvero lieto di confermare di aver firmato il decreto con cui è disciplinata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, che è ora in corso di pubblicazione. Vorrei precisare che questo provvedimento giunge in esito ad un percorso molto complesso che abbiamo concluso in tempi davvero ristretti, scongiurando la prospettiva, che aveva giustamente preoccupato i tantissimi aspiranti a queste graduatorie, di una mera proroga delle graduatorie precedenti. Ricordo infatti che il provvedimento recepisce le innovazioni introdotte dal nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 in materia di ordinamento professionale del personale ATA, che è entrato in vigore solo a gennaio di quest'anno. Tra le novità, tutte molto rilevanti, segnalo l'introduzione del nuovo profilo professionale di operatore scolastico e dei nuovi titoli di studio per l'accesso ai singoli profili professionali. Così, tra i nuovi requisiti di accesso a tutti i profili professionali, fatta eccezione per quello di collaboratore scolastico, figura ora anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Nella consapevolezza che l'acquisizione di questo nuovo requisito non sarebbe stata agevole per i tanti candidati alla prima immissione in dette graduatorie, siamo anche intervenuti legislativamente, con un emendamento al decreto-legge milleproroghe, per consentire l'inserimento con riserva in tali graduatorie a chi fosse sprovvisto della nuova certificazione, dando il termine di un anno per conseguirla. Grazie all'imminente aggiornamento delle graduatorie, abbiamo così garantito la continuità del servizio nelle istituzioni scolastiche e consentito a tanti lavoratori di cambiare Provincia per avvicinarsi al proprio nucleo familiare e aggiornare il punteggio. Questo risultato, per nulla scontato in considerazione delle tante innovazioni contrattuali cui abbiamo dato attuazione in pochissimo tempo, conferma la particolare attenzione che stiamo riservando al personale ATA, sul quale stiamo investendo con una pluralità di interventi di sistema, sia in termini di riqualificazione professionale sia in termini retributivi e di organico, com'è dimostrato dagli interventi in via di finalizzazione in materia di posizioni economiche e progressioni di area, oltre che all'impegno (già mantenuto) di proroga dei contratti a tempo determinato per l'organico aggiuntivo.

entrata in vigore delle graduatorie di terza fascia dal 1° settembre 2024. Questa misura avrà un impatto significativo per il personale ATA, permettendo loro di aggiornare i punteggi delle graduatorie, un passo cruciale per migliorare le loro posizioni lavorative. Non si può non riconoscere che questo aggiornamento regolare delle graduatorie è fondamentale non solo per il benessere dei lavoratori, ma anche per garantire un efficiente funzionamento delle scuole, perché il personale ATA è una risorsa fondamentale e indispensabile per il loro corretto funzionamento. Non ci resta ora che attendere l'apertura delle funzioni previste per il 28 maggio. Voglio anche ricordare che si deve a questo Governo il merito di avere individuato una soluzione per assicurare alle scuole il supporto di personale ATA aggiuntivo in grado di accompagnarle nel percorso di attuazione sia delle azioni inerenti al PNRR, sia di quella di Agenda Sud. Proprio a tale scopo, infatti, sono stati predisposti più interventi normativi nel corso del 2023. Inoltre, nel recente decreto-legge di coesione sono stati stanziati 18 milioni di euro per la stipula di contratti fino al 15 giugno 2024 a favore di collaboratori scolastici già impegnati nello svolgimento di progetti nell'ambito del PNRR e di Agenda Sud. Sud. La ringraziamo, Ministro, per il suo costante impegno verso il settore dell'istruzione; ancora una volta, ha mantenuto le promesse fatte ai lavoratori e alle istituzioni scolastiche. Il suo intervento evidenzia un'ulteriore vittoria in favore di tutti coloro che operano nel settore educativo e formativo, che attendono con ansia le decisioni che influenzano direttamente le loro vite. Come politici, abbiamo il dovere di considerare queste figure professionali per il ruolo che svolgono quotidianamente nella comunità scolastica. La Lega è al suo fianco per una scuola inclusiva, incentrata sullo studente, ma anche sulla valorizzazione del personale scolastico e dei docenti.

nei giorni scorsi è stato reso pubblico il *focus* «Il PNRR per la scuola e l'università: a che punto siamo?», nato dalla collaborazione fra Fondazione Agnelli e Fondazione Astrid. Il *focus* avrebbe evidenziato un ritardo significativo nella spesa dei fondi assegnati dal PNRR al settore istruzione. infatti, su un totale di 20 miliardi di euro assegnati, sarebbero stati spesi solamente 3,3 miliardi, il che solleverebbe preoccupazioni sulla tempestività e sull'efficacia dell'utilizzo di queste risorse cruciali per il settore educativo educativo e scientifico. Inoltre, sempre secondo il rapporto, sembrerebbe che la rimodulazione del PNRR abbia modificato le tempistiche delle misure di investimento e in alcuni casi rivisto al ribasso le cifre. Il rapporto sostiene che anche le riforme più ambiziose, come quelle su formazione, orientamento e formazione tecnico-professionali, risulterebbero aver in parte modificato la loro sostanza e che la spesa effettivamente sostenuta si attesterebbe al 17 per cento circa degli stanziamenti. Pertanto, si chiede di sapere, onorevole Ministro, qual è lo stato di avanzamento dei progetti del PNRR per l'istruzione e come si pensi di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti e con la qualità adeguata.

circa il reale stato di avanzamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero. Lo studio a cui si fa riferimento ha riportato, infatti, dati parziali o comunque incompleti.

anche gli interventi di competenza del sistema universitario e della ricerca. Dunque il rapporto deve essere fatto con riferimento a 17 miliardi e non 20. I dati relativi alla spesa sono stati rapportati a un importo più elevato e inoltre non appaiono aggiornati, infatti rispetto all'importo di circa 17 miliardi la spesa erogata si attesta oltre 3,8 miliardi, dunque siamo al 21,6 per cento, ai quali si aggiungono ulteriori 609 milioni, in liquidazione proprio nel 2024. La percentuale sale quindi oggi al 24,4 per cento, dunque oltre la media degli altri interventi del PNRR. Ripeto, siamo oltre la media degli interventi del PNRR. Abbiamo raggiunto puntualmente tutti gli obiettivi e i *target* previsti, i quali, a dire il vero, costituiscono l'unico reale parametro per la valutazione dell'avanzamento del PNRR. Anche le complesse riforme previste sono state puntualmente rispettate con l'adozione di trentasei decreti attuativi in meno di un anno e con tutte le procedure di reclutamento dei docenti avviate nei tempi previsti. La stessa Commissione europea, in sede di revisione del Piano, ha apprezzato in particolare il lavoro svolto sull'edilizia scolastica, riconoscendo il nostro impegno nell'incremento complessivo di risorse statali pari a circa 820 milioni di euro, proprio a dimostrazione dell'avanzato livello di attuazione degli interventi. Non si può ritenere quindi che si siano abbassate le ambizioni del PNRR istruzione, o che si siano ridotti gli investimenti complessivi. Sugli asili nido, ad esempio, abbiamo appena adottato un nuovo piano asili di 734,9 milioni di euro di risorse non PNRR, cioè di risorse nostre. Sulle scuole nuove abbiamo avuto l'aggiudicazione di un numero di interventi addirittura superiore al *target* previsto dalla Commissione europea. Per quanto riguarda invece l'investimento sui divari territoriali e sul contrasto alla dispersione scolastica, il dato della spesa riportato nella ricerca era riferito a prima dell'avvio dell'anno scolastico, quindi è un dato errato. Ad oggi la situazione è molto diversa e i dati riferiti al numero di studenti coinvolti, attualmente 1.519.797 tra studentesse e studenti, per oltre 327.000 percorsi formativi, sono assolutamente in linea rispetto al *target* finale. Concludo confidando che l'illustrazione in questa sede dei dati reali e verificabili possa aiutarci a favorire una riflessione davvero seria e costruttiva, oltre che scevra di pregiudizi, sulla grande sfida che il PNRR sta offrendo non solo al settore dell'istruzione, ma all'intero Paese.

Non avevo dubbi sull'impegno e gli sforzi profusi. Non solo avete speso per ben 3,8 miliardi, oltre quelli in liquidazione nel 2024, ma avete anche impegnato risorse aggiuntive come il piano asili, imprimendo così alle politiche scolastiche e alle riforme legate al mondo della scuola un'accelerazione mai vista, con tempi certi e rapidi. La continua enfasi posta solo sulle criticità e sui supposti ritardi, solo attraverso dati forniti in maniera parziale o incompleti da alcuni centri studi, a fronte invece di tutti gli obiettivi ad oggi raggiunti, rischia di produrre una forte sfiducia nei confronti di migliaia di scuole, istituzioni ed enti che invece stanno lavorando per l'efficace e puntuale attuazione del PNRR. Signor Ministro, Fratelli d'Italia apprezza il lavoro che lei e tutto il Governo state svolgendo: un lavoro prezioso che dimostra come finalmente, dopo anni di incuria e abbandono, il sistema scolastico sia finalmente tornato al centro della crescita del Paese, integrato pienamente alla dimensione europea. Siamo convinti che lei, signor Ministro, seguirà i lavori con il massimo impegno e la massima competenza per ottenere una trasformazione del Paese che lascerà una preziosa eredità alle generazioni future: un nuovo sistema educativo che garantisca il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando

fosse abbastanza palese che una delle problematiche dell'Italia è proprio la mancanza di un *mix* energetico maturo. Da qui alcuni obiettivi che vengono dal *green new deal* europeo, i fondi del PNRR che abbiamo ottenuto e che impegnavano il nostro Paese a stanziare 130 gigawatt da fonti rinnovabili, di cui 80 da pannelli fotovoltaici.

l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito nella legge 2 febbraio 2024, n. 11, che ha previsto il raddoppio delle trattenute applicate da GSE per la copertura dei costi di gestione degli impianti fotovoltaici che beneficiano del conto energia, col chiaro intento di spingere gli operatori all'adesione ad un sistema collettivo, ma con chiaro effetto disincentivante per chi non volesse esercitare tale opzione. Su tutti l'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, cosiddetto decreto agricoltura, dove si è resa estremamente difficile e gravosa la collocazione di impianti fotovoltaici all'interno delle aree agricole. Per questo noi le chiediamo quali sono gli intendimenti del suo Ministero per sviluppo delle rinnovabili in generale e per venire incontro a chi vuole impiantare pannelli fotovoltaici nei campi agricoli.

in relazione al quesito posto dagli onorevoli interroganti, che ringrazio, si evidenzia che le due norme citate non pregiudicano gli impegni assunti dall'Italia a livello europeo, né tantomeno segnano un cambio di rotta rispetto a quello che è l'obiettivo di sviluppo delle rinnovabili. Il Governo, a partire dal suo insediamento, ha invero fatto tutto o molto nell'ottica di un tempestivo raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e verde, sia attraverso misure di carattere settoriale, sia mediante vari interventi di semplificazione procedimentale come leva ulteriore per lo sviluppo delle rinnovabili, destinate a trovare prossima sintesi nel decreto legislativo di attuazione dell'apposita delega prevista dalla legge di concorrenza, la legge n. Sulla prima norma citata, quella legata al raddoppio delle trattenute da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), riferibile esclusivamente ai pannelli fotovoltaici installati mediante il decreto ministeriale Conto Energia prima del 27 settembre 2020, si evidenzia che, trattandosi di una quota a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici a fine vita, è restituita al detentore laddove si è accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo di riferimento. Sulla seconda norma citata, quella del decreto-legge agricoltura, essa va letta nell'ottica di uno sviluppo ordinato degli impianti rinnovabili sul territorio nazionale, che insieme alle aree idonee che le Regioni stanno definendo e quindi devono poi individuare sul proprio territorio, potrà garantire una pianificazione regionale delle aree utili all'installazione di impianti necessari al raggiungimento di quanto previsto nel Piano nazionale integrato energia e clima, tra l'altro, con una distinzione tra i 75 e gli 85 gigawatt (75 come valore minimo del PNIEC e 80 quelli in ripartizione). In ogni caso, voglio evidenziare come gli obiettivi europei prefissati devono essere raggiunti secondo un oculato un oculato *mix* di tecnologie differenti, anche molto differenti fra loro, a cui potrà partecipare in chiave prospettica non solo il grande eolico *off-shore*, previsto dal decreto energia di qualche mese fa, ma anche l'energia nucleare come fonte ad emissioni zero, tema sul quale - com'è noto - sono in corso riflessioni e studi per una *road map* che porti al suo sviluppo.

né all'uno né all'altro. Ma, se non riusciamo neanche a mettere i pannelli fotovoltaici a terra, che è l'impianto più semplice esistente, figuriamoci se riusciamo a realizzare impianti così complessi, con interessi contrastanti. Lei sa benissimo, per esempio, che sul nucleare non siamo ancora riusciti a individuare il sito unico per i rifiuti radioattivi e che, in tutte le occasioni in cui qualcuno si fa avanti, ad esempio il sindaco di Trino Vercellese, poi

è che, con una norma così stringente sul fotovoltaico in agricoltura, le Regioni tal quale diranno che le aree agricole non sono idonee, con un grande nocumento per la comunità italiana, che deve invece vedere lo sviluppo delle energie rinnovabili, se vuole raggiungere minimamente quell'autosufficienza energetica che pensavo fosse un elemento scontato dopo la crisi energetica e di gas che abbiamo avuto a causa della guerra in Ucraina.

che risulta ormai fondamentale per accompagnare il comparto agricolo nel suo percorso verso una decarbonizzazione sostenibile. Si tratta, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'investimento per lo sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare. Lei sta seguendo questo tema con grande attenzione e, quindi, sarà importante la risposta che ci darà oggi. oggi. Con queste disposizioni si propone di sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano. Come sappiamo, il biometano si ottiene dal biogas generato a partire dagli scarti dei prodotti agroalimentari, dagli escrementi animali, dai residui delle colture agricole e forestali. Ci si propone ora, però, di migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti, riconvertendoli alla produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. L'obiettivo dovrebbe essere la produzione di almeno 2,3 miliardi di metri cubi di biometano entro la fine di giugno 2026. Il suo decreto ha il fine di promuovere l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, a beneficio quindi di tutti i cittadini. Semplificando, è previsto un sostegno all'investimento, pari al massimo al 40 per cento delle spese sostenute, ed è prevista una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano. Possono beneficiare degli incentivi gli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, agricoli o a rifiuti organici, e gli interventi di riconversione a biometano di impianti agricoli esistenti. Le chiediamo, gentile Ministro, quale sia l'andamento di questa importante misura da lei messa in campo, che noi di Forza Italia sosteniamo - come lei sa - in modo convinto nell'interesse degli agricoltori, che sono i primi custodi dell'ambiente, e nell'interesse chiaramente anche dei cittadini,

Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. In merito al quesito posto, giova premettere che, nel processo di diversificazione delle fonti di energia, svolge un ruolo strategico la produzione di biogas e biometano. Una maggiore diffusione degli impianti potrà contribuire ad aumentare l'efficienza energetica delle imprese agricole, abbassando i costi dell'energia e aumentando la resilienza nel prossimo futuro. Il biometano è fondamentale altresì per ridurre la dipendenza energetica e al contempo per decarbonizzare i trasporti e le industrie pesanti, in cui, non riuscendo in cui, non riuscendo ad elettrificare i consumi, la molecola verde e l'idrogeno sono le uniche alternative per poter decarbonizzare i processi produttivi. Pertanto, anche nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono stati previsti dei *target* di incremento della produzione di biometano al 2030, per raggiungere i 6 miliardi di metri cubi annui, circa il 10 per cento della stima di consumo di gas che si prevede al 2030. In relazione alla misura del PNRR citata dall'onorevole interrogante, lo scorso 10 maggio si è conclusa la terza procedura competitiva con ottimi risultati, anche grazie all'indicizzazione delle tariffe all'inflazione. Sono stati 132 i progetti ammessi a finanziamento per impianti di produzione nuovi o riconvertiti per una capacità produttiva pari a 58,119 58,119 *standard* metri cubi all'ora, con un tasso di emissione superiore al 95 progetti prevedono la riconversione di impianti agricoli esistenti, mentre i restanti 72 la costruzione di nuovi impianti a rifiuti organici o di impianti agricoli ordinari quelli a rifiuti organici e 61 quelli agricoli). All'esito delle tre procedure competitive già svolte, i progetti ammessi agli incentivi sono in totale 157, per una capacità produttiva pari a 71.950 *standard* metri cubi, che corrisponde a una producibilità annua di circa 630 milioni di *standard* metri cubi, pari oltre al 25 per che il PNRR prevede di raggiungere nel 2026. Segnalo infine che, sempre nell'ambito della misura del PNRR, sarà aperta a breve la quarta procedura competitiva, che si svolgerà dal 3 giugno

bene che siano stati rivisti i meccanismi per incentivare sia la riconversione degli impianti esistenti sia quelli nuovi a biometano: questo consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci si era dati, e non è poca cosa. Il risultato sarà un miglior utilizzo degli scarti agricoli e dei rifiuti organici per produrre energia pulita - come lei diceva - a tutto vantaggio dei nostri concittadini e dell'ambiente. È segno anche di un utilizzo puntuale delle risorse europee del PNRR, di cui le siamo grati.

*(M5S)*. Signor Ministro, con la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 il Governo Conte ha stanziato 200 milioni di euro per l'istituzione di un fondo denominato Fondo nazionale per il reddito energetico, destinato prioritariamente a famiglie in condizioni di disagio economico, con l'obiettivo di sostenere il loro autoconsumo di energia mediante l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Precedentemente alla suddetta delibera CIPE, il reddito energetico è stato oggetto anche di leggi regionali. La prima è stata la legge della Regione Puglia n. 42 del 9 agosto 2019, mia prima firma - all'epoca ero consigliere regionale - con la quale si prevedeva l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle abitazioni di persone disagiate come misura per alimentare centinaia di impianti a favore di altrettante famiglie, dimostrando così che questa misura era concreta e che il reddito energetico funzionava e poteva rappresentare da subito, soprattutto mediante l'energia solare, ampiamente disponibile in tutti i territori del nostro Paese, una misura per alimentare tutte le famiglie, ma anche le imprese, dal punto di vista sia economico sia ambientale. Nei primi giorni di questa legislatura, uno dei disegni di legge che tutti noi senatori del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto presentare proprio per estendere il reddito energetico a tutte le Regioni d'Italia è stato l'Atto Senato 334. Tale disegno di legge del MoVimento 5 Stelle sul reddito energetico nazionale è stato, in un primo momento, posto all'esame in Commissione ambiente. Successivamente è stato considerato superato, in data 8 agosto 2023, è stato pubblicato un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto proprio a disciplinare il Fondo nazionale del reddito energetico. Grazie appunto ai 200 milioni stanziati precedentemente dal Governo Conte 2, i nuclei familiari in condizioni di disagio economico potranno utilizzare l'energia prodotta per l'autoconsumo, abbattendo così i costi delle proprie bollette. L'articolo 3 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2023, al comma 1, lettere *b)* e *c),* prevede: la realizzazione di una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal reddito energetico nazionale e per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati. Inoltre, prevede la pubblicazione dei bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. Con il decreto ministeriale 8 agosto 2023, citato dall'interrogante nella sua relazione iniziale, è stato istituito il Fondo nazionale reddito energetico come misura destinata ad agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo al servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. In merito alle tempistiche di emanazione del regolamento del Fondo, volto a disciplinare l'operatività dello stesso, l'adozione dello stesso da parte del Dipartimento competente è prevista entro questa settimana. Il regolamento disciplina nel dettaglio i requisiti soggettivi degli utenti beneficiari e dei soggetti realizzatori degli impianti, nonché quelli specifici relativi agli impianti fotovoltaici, concernenti, ad esempio, i componenti di nuova realizzazione, i servizi accessori e di monitoraggio, la manutenzione nel corso della vita utile. Il regolamento definisce, altresì, la modalità di accesso ai contributi in conto capitale e le relative tempistiche di erogazione a seguito della connessione dell'impianto sul punto del consumo, nonché le modalità di funzionamento del Fondo di natura rotativa. Nella prima decade di giugno il GSE aprirà un portale per censire a livello territoriale i vari soggetti realizzatori, mentre, nella seconda metà di giugno, la sezione dedicata all'acquisizione della gestione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari. Si ritiene che, entro la fine di giugno 2024, la misura sarà completamente operativa con una dotazione di 100 milioni. Nel 2025 saranno resi disponibili ulteriori 100 milioni maggiorati dai proventi di vendita dell'energia prodotta e non autoconsumata, che il GSE acquista gratuitamente, valorizza sul mercato, riversando nelle casse del Fondo i relativi profitti. Signor Presidente, mi sia permesso di fare una considerazione finale che riguarda i tempi. Vi sono stati dei dubbi in merito all'eventuale necessità di notifica o meno in Commissione, e quindi con l'interlocuzione con la Commissione, che hanno consumato molti mesi.

io avevo presentato un'interrogazione e lei mi aveva dato dei tempi, che poi non sono stati rispettati. Infatti, ogni mese dovevano uscire i decreti attuativi sulle comunità energetiche e poi è passato un anno. Io mi auguro, dunque, di essere smentito e che i tempi che lei oggi ha citato siano effettivamente rispettati, anche perché si tratta di una misura fondamentale per il nostro Paese.

questo le chiedo di estendere questa misura anche alle imprese. E i cittadini beneficiano dell'autoconsumo, cioè tutta l'energia che riescono a consumare è loro. L'energia invece in eccedenza, quella che non riescono a utilizzare, la valorizza lo Stato, alimentando così il Fondo. In questo modo ci guadagnano sia i cittadini sia lo Stato, con

tutti i tetti delle famiglie, delle imprese, i parcheggi, le barriere dell'autostrada e così via? Abbiamo delle superfici immense, già antropizzate, che possiamo utilizzare; dall'energia del sole, che è che è democratica e viene data a tutti i cittadini e a tutte le imprese ogni giorno, possiamo ricavare soldi sia per lo Stato che per i cittadini, senza andare a comprare energia fossile inquinante da Paesi spesso belligeranti. Mi auguro che ci sia veramente questo impegno e che i tempi siano rispettati, perché questa misura - noi abbiamo voluto da sempre, in Regione Puglia e anche con il Governo Conte, stanziando 200 milioni è solo all'inizio, ma secondo me ha delle potenzialità enormi, per cui è la prima misura da cui dobbiamo partire per solarizzare il nostro Paese.

Signor Ministro, vorrei porle alcune questioni molto importanti nei termini più semplici possibili. Dal 1980 al 2022 i disastri e le calamità naturali legati prevalentemente al cambiamento climatico hanno prodotto nel nostro Paese oltre 100 miliardi di danni. Negli ultimi dodici-ventiquattro mesi noi abbiamo avuto fenomeni estremi che hanno colpito, procedendo a ritroso e partendo dal più recente, la Lombardia e il Veneto in questa settimana e nella scorsa, a novembre 2022 la Toscana, nell'estate del 2024 nuovamente l'Emilia-Romagna, nel 2023 l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana. A fronte di questi eventi noi abbiamo dovuto registrare una decisione - a nostro avviso sconcertante - volta a tagliare i fondi destinati alla lotta al rischio idrogeologico nel PNRR del 51,7 per cento. Lo stanziamento originario era di 2,49 miliardi, lo stanziamento attuale è di 1,287 miliardi, con un calo di La disponibilità attuale è di 1,203 miliardi, molto meno della metà dello stanziamento originario. Questa decisione già di per sé è grave, ma più grave ancora sono le notizie che ci giungono dai territori. Io vengo dalla Toscana e posso dire dire quello che avviene in Toscana, ma in Lombardia, in Veneto, nelle Marche e in Emilia-Romagna, soprattutto, non accadono cose diverse. In Toscana noi abbiamo visto la struttura commissariale, guidata dal Presidente della Regione, stilare un elenco molto preciso e accurato di danni, inviare le stime al Governo e sono successe due cose: o non è successo niente oppure si sono fatte passerelle che hanno compreso la firma di decreti, che però poi si è scoperto essere del tutto inattuabili. Da noi il ministro Giorgetti ha fatto vedere che firmava un decreto di 67 milioni per la Toscana, ma debbo dare la notizia che quei soldi è come se non esistessero perché non si possono spendere, mancando i provvedimenti attuativi. Non si sa quando essi arriveranno e, quindi, ai cittadini della Toscana non è arrivato ancora nelle tasche un centesimo. Questo incrementa il senso di solitudine della cittadinanza e fa aumentare il sentimento di rabbia. Noi non abbiamo bisogno di impegni di spesa e di stanziamenti: abbiamo bisogno di soldi che vengono effettivamente erogati e questo non sta accadendo in nessuna delle Regioni colpite; o sta accadendo in misura molto limitata, per quanto riguarda non soltanto gli indennizzi ai cittadini, ma anche le risorse che servono alle strutture pubbliche per ripristinare le infrastrutture che sono state colpite dai disastri naturali. Solo in Toscana - cito di nuovo la Toscana perché la conosco meglio, ma non c'è una situazione diversa nelle altre Regioni - abbiamo avuto un fabbisogno di 1,2 miliardi per fare casse d'espansione, ripristinare alvei di fiumi, strade e ponti, ma non abbiamo ancora avuto niente. Io penso che questo ritardo sia davvero molto colpevole, che si debba passare dalle parole ai fatti, dagli stanziamenti alle erogazioni effettive e dal niente nelle tasche dei cittadini e delle imprese a qualcosa di concreto nelle tasche dei cittadini e delle imprese.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. In merito al quesito relativo alla eliminazione dal PNRR della misura relativa alla riduzione del rischio idrogeologico, la cui titolarità era attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si rappresenta che non si è verificato alcun definanziamento di interventi né rallentamenti, in quanto le risorse previste, pari a 1,287 miliardi di euro, erano state destinate esclusivamente ad interventi in essere, ovvero facenti parte di programmazioni già definite, alimentate da linee di finanziamento preesistenti rispetto al PNRR e che sono proseguite, anche perché opere in corso. inoltre come nella programmazione del piano stralcio 2024-2026 il MASE ha messo a disposizione delle Regioni e delle Province autonome complessivamente circa un miliardo di euro di risorse di bilancio e altre cospicue risorse sul tema del dissesto saranno previste a valere sulla programmazione e la coesione. In merito agli altri quesiti posti, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento della protezione civile, competente per materia, si evidenzia, in relazione all'alluvione del 15 maggio scorso sul territorio lombardo, che in assenza di una richiesta di deliberazione dello stato di emergenza da parte della Regione, il Dipartimento della protezione civile sotto il profilo operativo ha assicurato il costante monitoraggio degli eventi in stato di presidio operativo coordinando periodici punti di confronto con i territori interessati. In relazione alle risorse erogate per l'alluvione in Toscana, a seguito dello stato di emergenza, sono stati inizialmente previsti stanziamenti complessivi per 33,7 milioni. Nel Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024 (quindi (quindi meno di un mese fa) è stata deliberata un'ulteriore integrazione di 88,5 milioni, mentre il decreto-legge n. 39 del 2024 ha stanziato ulteriori risorse per 66 milioni di euro in favore dei privati e delle attività produttive, disponibili rapidamente sulla contabilità speciale del Commissario. Si tratta, quindi, di una valutazione che va fatta e in questo in questo senso possiamo anche sollecitare e verificare nuovamente. Riguardo all'alluvione in Emilia Romagna, il Dipartimento della protezione civile ha adottato una procedura sperimentale innovativa, per l'immediato sostegno ai soggetti privati per i danni subiti dalle abitazioni di primaria residenza. Ad oggi risultano liquidati circa 71 milioni per gli acconti e circa 32 milioni per i saldi, per un importo complessivo di 103 milioni di euro, di cui nove già nella prima decade di luglio 2023, a meno di due mesi dalla conclusione dei fenomeni alluvionali. Con riguardo ai tempi necessari per il riconoscimento dei ristori, il Dipartimento rappresenta che è allo studio apposito provvedimento con cui dare corso alle procedure per la concessione di contributi a favore di privati e imprese danneggiate dall'emergenza verificatasi negli anni 2022 ad eccezione di quelle per le quali sono intervenuti provvedimenti normativi di natura primaria. soddisfatti dalla sua risposta. Non più tardi di due giorni fa il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha raccontato come non siano arrivati assolutamente finanziamenti per coprire i beni mobili

insieme ai due giovani sindaci, e hanno spalato, cercando di mettere in sicurezza il territorio, ma c'è un problema grande come una casa: mancano le vasche di laminazione, che sono di competenza della Regione; magari potrebbero arrivare dei fondi, visto che siete voi ad amministrare la Regione Lombardia. Il problema è problema è che quando si fanno le vasche di laminazione, le si fanno in ritardo e noi non possiamo aspettare che queste vasche arrivino ora, quando è esondato il Naviglio della Martesana, che non è mai esondato nella storia. Di fronte ad una vera crisi climatica, sono necessarie misure straordinarie, per cui chiediamo un impegno chiaro affinché quei fondi arrivino nel più breve tempo possibile, affinché la vasca di laminazione lì venga realizzata nel più breve tempo possibile e arrivi il sostegno a queste famiglie. Il sindaco di Bellinzago Lombardo ha dormito con gli sfollati negli scorsi giorni; sono stati tutti accolti nella scuola media del territorio, sono rimasti senza casa come è accaduto a tantissimi cittadini italiani nel corso degli ultimi due anni. Abbiamo bisogno di un Governo che dica in maniera estremamente chiara che sa

Da quest'Aula mandiamo un abbraccio a tutti i sindaci e a tutte le popolazioni che sono state colpite da questi eventi gravissimi. A nessuno sarà sfuggito come proprio in quei Comuni siano stati tratti in salvo dagli asili nido dei bambini da due carabinieri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

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Napoli è una città ricca di fascino e di storia, con tanti tesori nascosti e segreti da svelare. Tra le meraviglie più affascinanti e forse meno conosciute della città c'è la Galleria borbonica, un complesso sotterraneo che racconta le vicende e disvela l'aspetto più romantico della città partenopea. La storia di questo luogo è avvincente e ricca di mistero, in quanto ha svolto diverse funzioni nel corso dei secoli, dalle antiche cave di tufo alla sua utilizzazione come rifugio durante la Seconda guerra mondiale. Ebbene, ho avuto il piacere di esplorare questo sito meraviglioso, che trae origine dall'ingegno borbonico ed è stato riportato all'antico splendore attraverso un'importante ed intelligente opera di bonifica a proprie spese dei fratelli Luca e Marco Minin. È indubbio che i due fratelli vanno supportati, per sostenere e valorizzare l'importante impegno a vantaggio di tutta la collettività. È compito però dello Stato supportare ed affiancare tutti gli speleologi e geologi come loro, che negli ultimi decenni hanno ricostruito la Napoli del sottosuolo, a partire dal celebre Ulisse Lapegna, che ha avuto il merito di mappare minuziosamente le cavità partenopee. Tuttavia, onorevoli colleghi, in pochi sanno che il ventre di Napoli accoglie anche una gigantesca discarica che potrebbe sfiorare il mezzo milione di metri cubi di spazzatura, come mi hanno spiegato i gestori della Galleria borbonica e come ho potuto constatare di persona. Con mia somma meraviglia, direi rammarico, ho sperimentate di che cosa è capace l'uomo. C'è un ammasso di rifiuti stratificato nel tempo che è stato smaltito nei decenni attraverso gli antichi pozzi, ancora oggi presenti nella maggior parte dei palazzi del centro storico di Napoli. Si è così alimentata una discarica che esprime l'aspetto più oscuro delle nefandezze nascoste nelle viscere della terra. Oltre al materiale inerte depositato già durante la seconda guerra mondiale, sono state ritrovate anche cumuli di materiale pericoloso, come agenti chimici e grandi quantità di amianto: una bomba ad orologeria che non può essere ignorata. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi a questo quadro a tinte fosche, i Ministeri competenti hanno il dovere di agire per tutelare la salute dei napoletani, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. Eppure non sembrano esserci progetti concreti per bonificare il nostro sottosuolo. Certo, non è un'operazione semplice né a costo zero, ma è chiaro che necessita di una disponibilità di fondi per progettare la rimozione di milioni di metri cubi di rifiuti di tipo vario attraverso i pozzi. Tenuto conto che gli sversamenti continuano ancora a tutt'oggi, si impone di individuare e di studiare meccanismi per interrompere questo malcostume che si realizza e che continua ad alimentare illecitamente l'accumulo dei rifiuti attraverso i pozzi presenti negli edifici. A tal proposito, sposo in pieno la proposta di Gianluca Minin, considerato un luminare del sottosuolo in Italia, secondo cui andrebbe imposta ai condomini, soggetti responsabili che vivono sopra le discariche, di occuparsi a loro spese della rimozione; la trovo una scelta razionale e positiva. Ma ciò implica l'accertamento, perciò è compito dello Stato determinare un nesso di causalità e di responsabilità,

confluissero in un fondo per valorizzare il sottosuolo e per manutenere il sito. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è arrivato il momento di alzare il tappeto di rifiuti che ristagna, per far rivivere la bellezza delle cavità sotterranee e realizzare i versi della canzone di Pino

il 23 maggio 1992 una strage terroristica mafiosa uccise il giudice Giovanni Falcone, la magistrata e moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. Ci furono 23 feriti. Chi è Giovanni Falcone? Magistrato infaticabile e capace di intuizioni geniali, come quella di seguire i soldi per cogliere e comprendere le dinamiche criminali, quello che sarà poi chiamato il "metodo Falcone". Il 21 giugno 1989, 500 candelotti di tritolo vengono scoperti sugli scogli dell'Addaura, nei pressi della villa dove soggiornava Falcone. Quel fallito attentato turba molto Giovanni Falcone, che parla di «menti raffinatissime». Il 23 maggio a Capaci la strage avviene alle 17,58: le tre auto sono all'altezza dello svincolo di Capaci e in quel preciso istante Giovanni Brusca, appartato sulla collina, accanto all'autostrada A29, aziona il telecomando che fa esplodere 1.000 chili di tritolo. L'autostrada si frantuma, è una scena apocalittica. L'Italia è sconvolta da quella violenza inaudita; è una delle pagine più strazianti della storia italiana. La vicenda giudiziaria porta alle condanne di tutti i vertici di cosa nostra, ma ancora la verità processuale non è stata tutta scritta. Ci si domanda ancora se i vertici di cosa nostra l'abbiano fatta da soli. Tanti depistaggi, coperture, collusioni e connivenze ci dicono che ancora non conosciamo pienamente la verità. Chi era Francesca Morvillo? Francesca, bravissima magistrata, anche del tribunale per i minorenni, non è morta solo perché era la moglie di Giovanni Falcone, ma perché, come lui, aveva fatto una scelta precisa, quella di stare accanto a Giovanni, ma contro le mafie e contro le organizzazioni criminali. Francesca si era cibata di diritto e codici, un tratto che ha caratterizzato sempre la sua personalità, il suo lavoro: una grande sensibilità e una profonda umanità. Il 23 maggio 1992 era accanto a Giovanni. Chi è Rocco Dicillo? Nasce a Triggiano in provincia di Bari. Aveva un naturale senso di giustizia, orgoglioso di fare parte della scorta del giudice Falcone; un uomo pieno di progetti e passione. La sua fidanzata Alba disse di lui: «Rocco non era soltanto un uomo della scorta, Rocco era un uomo di trent'anni anni che aveva aspettative di vita, come tutti quanti noi. Lui mi diceva sempre: Alba, troverai sempre una risposta nella nostra Costituzione». Il 23 maggio, in quel caldo sabato, era accanto al suo giudice. Chi è Antonio Montinaro? Non era solo il caposcorta, ma era un giovane, un marito, un padre. Nasce a Calimera, provincia di Lecce, in una famiglia nella quale ci si nutriva di pane, Bibbia e Costituzione. Lavora con professionalità, dedizione, spiccate qualità professionali e morali. Voglio ricordarlo con le sue parole: «Chiunque fa questo lavoro ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. (...) Io, come tutti gli uomini, ho paura indubbiamente, ma non sono un vigliacco». Il 23 maggio era accanto a Giovanni Falcone. Chi è Vito Schifani? Poliziotto, atleta, padre, marito, un giovane pieno di sogni; nasce a Palermo, si arruola nella Polizia, il suo alto senso dello Stato e delle istituzioni lo portano a questa scelta di vita, che assolve con profonda dedizione e responsabilità. Il 23 maggio era accanto a Giovanni Falcone. Oggi nella Giornata della legalità li vogliamo ricordare. Il loro coraggio e il loro senso di giustizia è un bene che appartiene al Paese e a tutti noi. *(Applausi)*. **Atti